il 21 dicembre 2005 è stata promulgata una norma, su proposta dell'allora senatore Calderoli, che riformava la legge elettorale. Quella norma è diventata poi famosa perché lo stesso stesso ministro Calderoli la definì una "porcata", divenendo così nota come *porcellum*. Siccome abbiamo a cuore il senatore e ministro Calderoli, a cui ci lega un profondo rispetto e affetto, per evitare che anche l'autonomia differenziata diventi un'altra porcheria, visto quanto pubblicato ieri dal Servizio del bilancio Senato, chiediamo un'informativa urgente da parte del Ministro per chiarire gli aspetti che detto Ufficio ha evidenziato e che trovano il Gruppo MoVimento 5 Stelle totalmente d'accordo. Con questo intervento chiediamo pertanto un'informativa urgente, il prima possibile, del ministro Calderoli sul tema.

loro vicini e faremo tutto il possibile per aiutare e sostenere gli sforzi della Protezione civile, delle istituzioni regionali, dei sindaci, degli amministratori che si stanno spendendo in queste ore, senza sosta, per dare sollievo. Il nostro è un Paese fragile, bisognoso di grande unità in questi momenti e sono sicuro che il Governo, insieme alla Regione, sapranno dare risposte adeguate con tutto il nostro sostegno. Per ora, esprimiamo davvero la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, la nostra attiva presenza nei confronti di tutti coloro che stanno soffrendo e a cui il Senato si sente vicino.

Presidente, vorrei associarmi alle dichiarazioni di espressione della massima solidarietà da parte del nostro Gruppo alle popolazioni colpite, ai Presidenti delle Regioni, che stanno facendo il loro dovere in questo momento, ai tanti sindaci coinvolti. Sono momenti di dolore che però non possono in alcun modo non indurci ad avere un atteggiamento molto serio di programmazione per il futuro. Come le è noto, signor Presidente, noi abbiamo chiesto ripetutamente al Governo e al Parlamento di fare il punto sulla necessità di ripristinare l'unità tecnica di missione ItaliaSicura per la lotta al dissesto idrogeologico. la richiesta di un'informativa urgente della Presidente del consiglio, che abbiamo chiesto anche per iscritto alla Presidenza, perché

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia

Se la votazione è per alzata di mano qualcuno deve anche guardare, osservare. I Gruppi possono anche chiedere la votazione elettronica quando lo ritengano, altrimenti non ci sarebbe la differenza tra la votazione per alzata di mano e la votazione elettronica, senatore Magni.

Dico inoltre al senatore Magni che avevo visto bene le mani alzate, perché chi presiede ha anche il compito di intuire quali voti sono di più e quali di meno; si può sbagliare e la controprova esiste a garanzia della volontà dell'Assemblea. Quindi seguiamo le regole, compresa la stima delle mani

Nonostante riteniamo condivisibile, infatti, la *ratio* del provvedimento, a nostro parere si doveva fare qualcosa di più. La cosiddetta riforma Cartabia del processo penale, penale, con l'obiettivo di ridurre il numero dei procedimenti giudiziari, quindi con una finalità deflattiva, ha ampliato il catalogo dei reati per i quali la procedibilità è subordinata alla presentazione di querela da parte della persona offesa. Da lì sono emerse delle criticità che hanno reso doveroso un intervento normativo *ad hoc*, quello presente. In particolare, a destare l'allarme non sono stati solo gli operatori del settore, ma anche autorevoli esponenti dell'attuale maggioranza di Governo e del Governo stesso, che hanno definito la riforma addirittura un disastro e hanno annunciato un intervento di forte discontinuità. In realtà, almeno stavolta non è stata scelta la decretazione di urgenza, ma un intervento "chirurgico", attraverso un disegno di legge, scelta che noi condividiamo. Ad esempio, i reati procedibili a querela diventano procedibili d'ufficio se ricorre l'aggravante del cosiddetto metodo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis*, primo comma, del codice penale, la stessa valutazione è stata compiuta anche rispetto ai reati connotati dall'aggravante della finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-*bis*, primo comma, del codice penale. In entrambi i casi, il provvedimento di cui si tratta interviene apportando proprio dei correttivi. Inoltre, è stata introdotta una correzione del codice antimafia, prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per le lesioni personali e l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, per il quale è necessario che le Forze dell'ordine e di polizia che intervengono si adoperino per ottenere la querela della persona offesa, se non è presente sul luogo del reato, nelle quarantott'ore successive. Oltre a questi casi, in cui l'intervento del Parlamento è certamente opportuno, la prassi applicativa ha immediatamente evidenziato altre criticità in altri ambiti, sui quali però si è deciso - sbagliando a nostro parere - di non intervenire. Secondo noi, infatti, avremmo potuto fare qualche sforzo in più, approvando emendamenti che però hanno avuto tutti parere contrario e poi sono stati bocciati. Di conseguenza, come detto in premessa, non possiamo esprimere un voto favorevole, per quanto correttamente sia stata confermata l'impostazione della riforma e per quanto correttamente lo strumento utilizzato, quello del disegno di legge, abbia portato all'attenzione dell'Aula correttivi ragionevoli. Il rifiuto di ogni contributo offerto dalle opposizioni, anche su temi molto sensibili, estremamente delicati e crediamo condivisibili, ci impone dunque l'astensione.

oggi, in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, dimostra una capacità da parte dello Stato - in questo probabilmente un Esecutivo può fare

nello sviluppo di quello che può essere il processo di carattere penale, soprattutto andando a difendere quelle persone che vivono in contesti particolari. *(Brusio)*. Vi

Prego, senatore Salvitti.

quindi di un intervento puntuale, preciso e pragmatico che va ad incidere chirurgicamente sul quadro normativo attuale per permettere agli inquirenti un

dà un effettivo sostegno, soprattutto alla parte inquirente, al di là del procedimento di carattere penale. Esso non incide solamente su questo, ma anche sulla flagranza di reato,

apparire minori. Questa è la dimostrazione di un'attenzione particolare e soprattutto della velocità di intervento da parte di un Esecutivo che dà la possibilità di agire con maggiore tranquillità e con maggiore velocità soprattutto su reati che

Devo cominciare con un plauso al Governo dal punto di vista tecnico- procedurale, perché sicuramente abbiamo apprezzato il fatto che l'annunciato decreto-legge non è stato adottato; il Governo ha deciso per un disegno di legge che chirurgicamente va a sistemare sicuramente due falle che si erano prodotte a seguito della delega Cartabia e dell'assunzione dei decreti delegati. Quindi, per i reati

di reato. Voglio dire in premessa che la riforma Cartabia è stata un'ottima riforma, innanzi tutto per il metodo con il quale è stata adottata. Ricordiamo che non è stata probabilmente la riforma ideale per nessuno, però è stato un faticoso esercizio di raggiungimento di un equilibrio, per il quale credo che quest'Aula debba anche esprimere un ringraziamento all'ex ministra Cartabia che si è molto spesa e ha portato a casa una riforma importante - ricordiamolo - anche per i fondi del PNRR, perché ci muoviamo sempre in quest'ottica. Va detto anche che la bontà della riforma è dovuta anche all'idea che più reati vengano perseguiti a querela piuttosto che d'ufficio.

lo Stato decide che un reato è perseguibile a querela di parte è perché fondamentalmente se ne lava le mani, lascia alle parti. Ma io non penso che sia così. Nel momento in cui lo Stato stabilisce che c'è una sanzione penale,

viene investito delle sue caratteristiche di reato, di crimine, è di per sé un fatto che ha una rilevanza pubblica. Che poi quella rilevanza pubblica venga esercitata o meno, a seconda che ci sia la querela o meno, ciò alla natura pubblicistica dell'intervento dello Stato. Altrimenti dovremmo immaginare la sanzione penale come una sorta di clava che viene messa in mano alle parti,

alle vittime un'arma per vendicarsi dell'autore del reato. Una visione del diritto penale di questo genere, secondo me, va rigettata alla radice: qualsiasi reato, che sia procedibile a querela di parte o d'ufficio, ha rilevanza pubblica, perché il giudice il giudice decide quella sanzione in nome del popolo italiano. Detto questo, non tutti i reati possono essere perseguibili d'ufficio, perché non è che lo Stato si può occupare di tutto. Noi lavoriamo e e viviamo in un ordinamento in cui è prevista l'obbligatorietà dell'azione penale, pertanto le azioni penali ricadono sulle procure, che devono occuparsi di tutto. C'è un emendamento della collega Lopreiato che vuole reintrodurre la procedibilità d'ufficio, se la violazione di domicilio viene fatta attraverso una violenza sulle cose: se io rompo una maniglia per entrare in una proprietà privata, c'è una violenza sulle cose, quindi la procedibilità d'ufficio. Diventa difficile esercitare l'obbligatorietà dell'azione penale, se tutto dev'essere procedibile d'ufficio. l'ex ministra Cartabia e bene abbiamo fatto noi a cercare di deflazionare, introducendo il principio che la querela di parte dev'essere più utilizzata. Aggiungo un altro motivo:

c'è l'arresto in flagranza, se la persona offesa non è prontamente reperibile, scatta la privazione della libertà personale. viene alla luce l'idiosincrasia di questo Governo con il concetto di libertà personale. Voi ci state abituando a questa sorta di fabbrica del reato tale per cui in Commissione ormai ci guardiamo quasi sorridendo (se non ci fosse da disperarsi), pensando è arrivato il reato della settimana (ogni giorno ce n'è uno: oggi si parlava di di *baby gang*, siamo curiosi di sapere cosa volete fare della giustizia minorile). Cosa decidete, dunque? Che una persona, arrestata in flagranza per un reato per il quale non esiste la procedibilità d'ufficio, dev'essere privata della libertà personale. Addirittura, viene sospeso il processo per direttissima nell'attesa di trovare il querelante. Cari signori

di andare a trovare una persona offesa che è talmente interessata dall'offesa da essere irreperibile. Ma siamo seri! È chiaro che, messo tutto insieme, ci troviamo davanti alla riparazione di un problema, perché è ovvio che, se c'è un reato mafioso o di stampo terroristico, è giusto che ci sia la procedibilità d'ufficio. Il resto di questo disegno di legge, però, francamente non si regge in piedi ed è anche preoccupante, appunto perché esprime una cultura

che non si può davvero vedere. Di conseguenza, messe insieme una valutazione molto positiva sull'articolo 1 e una posizione molto negativa sull'articolo 3, mi sembra che la cosa più logica e coerente da fare, da parte del nostro Gruppo, sia quella di astenersi. E così faremo. *(Applausi)*.

Il Gruppo, infatti, condivide tutte le considerazioni da lui svolte in modo dettagliato sull'articolato in esame. Il disegno di legge del ministro Nordio, come ben sappiamo, nasce dalla necessità di rivedere alcuni aspetti della cosiddetta riforma Cartabia, che abbiamo condiviso e condividiamo. Con tale riforma, appunto, aumentano i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa. Oggi votiamo il testo così come modificato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione giustizia del Senato non ha ritenuto, giustamente, di apportare ulteriori variazioni. Le modifiche sostanziali introdotte alla riforma Cartabia prevedono ora la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del metodo mafioso, ma anche per quelli che hanno finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Quest'ultima circostanza, in particolare, si evidenzia appropriata, in relazione alla recrudescenza dei fenomeni legati alla galassia anarchica, e non solo, sui quali ci sono un'allerta puntuale ed un monitoraggio delle Forze dell'ordine. Viene inoltre modificato il codice antimafia, prevedendo ora la procedibilità d'ufficio per il reato di lesione personale, quando è commesso da una persona sottoposta a una misura di prevenzione personale fino ai tre anni che seguono il termine di tale misura. La Camera ha quindi introdotto le giuste modifiche, posto che risultava evidentemente irragionevole il fatto che nell'elenco dei reati per i quali era prevista la procedibilità ci fossero i delitti di violenza privata e minacce, mentre fosse escluso il delitto di lesione personale. L'altro ramo del Parlamento ha inoltre modificato la disciplina del giudizio direttissimo, che viene ora coordinata con le nuove disposizioni in materia di arresto in flagranza, obbligatorio per i delitti procedibili a querela. Con le modificazioni inserite, il giudice dovrà sospendere il processo ove manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima di questo. Insomma, si pone rimedio alle criticità riscontrate in sede di applicazione della nuova normativa della riforma Cartabia alle ulteriori problematiche a questa correlate, che hanno tra l'altro animato il dibattito in quest'ultimo anno, fuori e dentro le aule parlamentari. Riscontrate dunque in sede di esame del disegno di legge in Parlamento queste criticità, si è agito. Bene ha fatto il Governo a sostenere quest'azione e bene ha fatto il Parlamento, nei suoi due rami, ad approvare tale testo.

annuncio il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle, perché il testo di legge, così come formulato, si limita a porre rimedio a una delle più gravi storture della riforma Cartabia, ma ne lascia sussistere altre, di analoga gravità, che sarebbe stato possibile eliminare, se fossero state accolti, in tutto o in parte, i nostri emendamenti. storture sono state determinate dalle scelte politiche discrezionali che sono state operate dal Governo Draghi, che ha elaborato i contenuti precettivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. scelte politiche discrezionali hanno di molto travalicato, in più punti qualificanti, la *ratio* della delega legislativa ricevuta dal Parlamento con la legge del 27 settembre 2021, n. 134, che proprio per questo motivo non sono state condivise dal MoVimento 5 Stelle, come risulta da parere contrario espresso nella seduta del 15 settembre 2022 della Commissione giustizia allo schema di decreto legislativo che ho citato. Quali fossero la *ratio* della legge delega e la volontà del Parlamento risulta in modo inequivocabile dalla stessa relazione illustrativa

«La legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilità a querela in rapporto a reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali». E ancora: «Si è pertanto conservata la procedibilità d'ufficio

per rendersi conto come questo brano della relazione illustrativa sia una pubblica ammissione da parte del Governo di avere platealmente travalicato i limiti della delega legislativa, operando la scelta di declassare al rango di reati procedibili a querela anche reati gravi, come il sequestro di persona, nei quali è contestata l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo o di eversione, tenuto conto che la dimensione sovra-individuale, la particolare gravità di tali reati e lo stato di soggezione delle vittime sono fatti notori e di tale palmare evidenza da non richiedere alcuna illustrazione. Quello che è grave è che tale declassamento non è stata un'imperfezione dovuta a un *deficit* di attenzione di un legislatore frettoloso; quel declassamento è piuttosto la spia, il momento di emersione e di massima visibilità dell'ideologia che, dietro il velo di un neutrale tecnicismo, ispirato solo da ragioni di efficienza e di razionalizzazione delle risorse, attraversa, come un fiume carsico sotterraneo, altri aspetti fondamentali della riforma Cartabia, che ha ispirato anche la scelta di declassare a reati procedibili a querela, unitamente a quelli di mafia, anche altri gravi, lesivi di beni di rilevanza costituzionale, quali l'integrità e la libertà personali. Per darvi contezza della gravità delle scelte politiche operate al riguardo dal Governo Draghi col decreto legislativo che ho citato, mi limito a un solo esempio. Un pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, dichiarato delinquente professionale, sfonda a spallate e calci la porta di un'abitazione privata, aggredisce e pesta a sangue il proprietario e la moglie, provocando loro lesioni giudicate guaribili sino a quaranta giorni, distrugge il mobilio dell'abitazione e sega tutti gli alberi del giardino, tiene sotto sequestro i due coniugi per due settimane, adoperando sevizie e agendo con crudeltà verso i sequestrati. Ebbene, nel film dell'orrore che vi ho appena esemplificato, la data del 10 ottobre 2022, nella quale è stato approvato il decreto attuativo della riforma Cartabia, segna uno spartiacque storico nel rapporto Stato-cittadino. Prima di tale data, tutti i reati consumati nella sequenza che ho descritto erano perseguibili d'ufficio e ve li specifico: reato di violazione di domicilio con violenza sulle cose; reato di lesioni personali con prognosi superiore a venti giorni e sino a quaranta giorni; sequestro di persona aggravata; danneggiamento con violenza della persona. Dopo quella data, tutti i reati indicati sono divenuti perseguibili a seguito di querela, perché - per ripetere testualmente le parole della relazione governativa citata - sono stati considerati «di non particolare gravità» e perché - testualmente - non «viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa». In altri termini, reati come il sequestro di persona ed altri ancora, che ledono beni di rilevanza costituzionale, sono stati considerati dal Governo non più eventi di rilevanza sociale e pubblica tali da imporre allo Stato di intervenire autonomamente, ma sono stati declassati a vicende interindividuali tra aggressore e vittima, che possono trovare un'autoregolazione transattiva, consentendo così di risparmiare risorse e tempo alla giustizia penale. Ci troviamo, in sostanza, dinanzi a: una profonda trasformazione del rapporto tra Stato e cittadino operata dal Governo Draghi; a uno strisciante ed occulto ridimensionamento del ruolo dello Stato nella società civile; a una trasformazione dello Stato da garante della sicurezza collettiva e tutore di beni individuali di rilevanza costituzionale in un ente prestatore di servizi a domanda, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio. Si tratta di una scelta politica del Governo che costituisce una perfetta declinazione dell'ideologia politica neoliberista, divenuta ormai egemonica e senso comune, che da circa un trentennio è stata messa in opera per ridimensionare il ruolo dello Stato nella sanità pubblica, nella scuola pubblica e in altri settori fondamentali dello Stato sociale, che, dopo una lunga sperimentazione, ora viene applicata anche nel settore cruciale della giustizia penale. Si tagliano i costi della sanità tagliando la sanità, si tagliano i costi della giustizia tagliando la giustizia. *(Applausi)*. Una sorta di privatizzazione della giustizia penale, realizzata mediante un arretramento progressivo dello Stato nella regolazione dei rapporti sociali, al quale corrisponde una dilatazione progressiva dell'autoregolazione sociale, che imita l'autoregolazione del mercato. Un'ideologia, questa, della preminenza da accordare all'autoregolazione sociale, che viene applicata al sistema sociale sulla base di un presupposto teorico in larga misura falso, e cioè che nel conflitto sociale aggressore e vittime sono pariordinati, equipotenti e tutte le vittime sono sempre libere di autodeterminarsi e di scegliere se presentare querela o meno, optando per la soluzione che più soddisfa i propri interessi, così come qualsiasi operatore di mercato. Una falsità, questa *(Applausi)*, che è autoevidente, non solo per le vittime dei reati di mafia, ma anche nella vasta fenomenologia dei casi nei quali esiste un'asimmetria di rapporti di forza tra autori dei reati e parti offese e nei quali la vittima, pur non essendo incapace per età o per infermità, tuttavia, per fragilità di carattere, per lo stato di paura in cui versa o per il timore di subire ritorsioni, non si trova nelle condizioni di esercitare liberamente la scelta di presentare querela, lanciando così una sorta di guanto di sfida personale all'aggressore. In tutti questi casi, la scelta politica operata dalla riforma Cartabia di disattivare l'intervento d'ufficio dello Stato a tutela delle vittime appare criminogena, perché si risolve nell'abbandono dei fragili e in un premio ai violenti. Una scelta politica tanto più irragionevole, ove si consideri che la stessa riforma Cartabia ha previsto all'articolo 152 del codice penale che non è valida la remissione tacita della querela, quando si accerti che la parte offesa versa in uno stato di particolare vulnerabilità, che può essere desunta, ai sensi dell'articolo 94-*ter* del codice procedura penale, dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Vi sembra razionale ammettere, per un verso, che la parte offesa possa non essere libera di autodeterminarsi quando rimette la querela, perché particolarmente vulnerabile e, nello stesso tempo, sostenere invece che è sempre libera di autodeterminarsi, quando deve presentare la querela, e che quindi è giusto *(Applausi)* prevedere che reati gravi come il sequestro di persona possano essere perseguiti solo a seguito di querela? Erano altre le strade da seguire per deflazionare il carico penale senza compromettere diritti essenziali. Invece di procedere con il bisturi chirurgico, si è usato il machete, senza equilibrio e misura. In conclusione, Presidente, per evitare di ratificare queste ed altre storture, avevamo avevamo presentato una serie di emendamenti, che sono stati rigettati senza alcuna spiegazione; ne prendiamo atto e insieme a noi ne prendano atto e ne serbino memoria i cittadini, ogni volta che subiranno violenza e sentiranno tutto il peso della loro fragilità e della loro solitudine, perché la maggioranza della classe politica di questo Paese ha deciso che è cosa buona e giusta che lo Stato abbandoni al proprio destino i fragili e le persone vulnerabili per tagliare i tempi e i costi dell'amministrazione della giustizia.

Faccio riferimento anche all'intervento appena concluso dal collega Scarpinato. La riforma Cartabia è stata varata dal Governo Draghi e non dal Governo Meloni.

Si è intervenuti, con questa proposta del ministro della giustizia Carlo Nordio, approvando anche un procedimento d'urgenza per eliminare questo tipo

Storture e distorsioni in che senso? La cosiddetta riforma Cartabia ha portato a un ampliamento del novero dei reati procedibili a querela. Non mi dilungo sull'illustrazione del provvedimento, che è già stata fatta magistralmente dal relatore Zanettin, Zanettin, che ringraziamo anche per l'equilibrio dimostrato e per la grande virtù che ha l'avvocato e il giurista, ossia la prudenza. Ringrazio anche tutta la Commissione giustizia, perché su questo tema credo che abbiamo avuto alcune convergenze, tant'è che mi sorprende l'ultimo intervento del collega del MoVimento 5 Stelle. Il disegno di legge in esame va ad intervenire su ipotesi

proposta una modifica per far sì che, in presenza dell'aggravante mafiosa o per terrorismo, il reato sia sempre procedibile d'ufficio.

Si interviene poi a colmare una lacuna del codice antimafia, dal quale, forse non ragionevolmente, era stato eliminato il reato di lesione personale. Oggi invece, con questa modifica, il reato di lesione personale diventa sempre procedibile d'ufficio, quando è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale

perché è una decisione che viene presa direttamente dal Governo e dal Parlamento, escludendo alcuni reati e delitti e trasformandoli magari in contravvenzioni, oppure declassandoli a sanzioni amministrative.

Queste scelte sono state fatte a suo tempo per affrontare varie tematiche, *in primis* il sovraffollamento carcerario e la spada di Damocle della sentenza Torreggiani. Con la ministra Cartabia si è fatta una scelta, perché occorreva rispondere

i tempi con una riforma che ha valorizzato la procedibilità a querela. Si è inserita la riforma all'interno degli obiettivi del PNRR, dicendo che per noi l'efficienza, per rispondere alle richieste e ottenere i fondi del PNRR, significava arrivare a una riduzione dei tempi, diminuendo il numero dei procedimenti con la remissione della querela, con con l'esclusione di molti reati dalla procedibilità d'ufficio e assoggettandoli invece a una procedibilità a querela. Tuttavia, tale realtà ha una caratteristica.

di questa importante riforma, eventualmente raccogliendo anche correttivi, come stiamo facendo ora su questo tema penale e come mi auguro faremo anche in campo civile, in cui ci sono difficoltà molto rappresentate che dai colleghi avvocati. parlando di una scelta che è stata adottata, perché la procedibilità a querela rimette nelle mani della persona offesa la scelta di procedere, quindi non gli fa passare sopra la testa la depenalizzazione o la scarcerazione del criminale, ma fa sì che sia la persona a

la seconda riguarda l'arresto in flagranza in assenza di querela nei reati procedibili a querela. Cito queste due questioni perché anzitutto mi sento di dover correggere le affermazioni che hanno fatto quasi tutti i colleghi, questo caso si interviene per correggere la riforma Cartabia: non è così. Qui si interviene per correggere alcuni princìpi che già esistevano prima della riforma Cartabia

sia per quanto riguarda la procedibilità a querela, considerando di introdurre la procedibilità d'ufficio per i reati per i quali ci sia l'aggravante del metodo mafioso,

Questo non si è mai fatto ed era un principio che non c'era nel nostro ordinamento. Ebbene, per un maggiore equilibrio tra le esigenze di tutela della persona offesa e le e le esigenze cautelari connesse all'arresto, abbiamo deciso di introdurre il principio per cui si può arrestare anche in assenza della querela presentata sul posto dalla persona offesa, salvo che la querela debba essere presentata nelle successive Noi condividiamo questi principi, che non mettono in discussione - lo voglio dire con grande chiarezza - le scelte che ha fatto la riforma Cartabia,

quasi all'unanimità, con l'eccezione certamente di Fratelli d'Italia, che allora era all'opposizione, ma tutti gli altri Gruppi parlamentari hanno votato a favore. Quella riforma riforma dava un principio di delega al Governo: trasformare in reati procedibili a querela quelli contro la persona e il patrimonio che avessero una pena minima edittale non superiore a due anni, anni, considerati quindi non particolarmente gravi. Questo era il principio di delega che abbiamo affidato al Governo quasi alla unanimità, con l'eccezione di Fratelli d'Italia. A questo principio si è attenuto il Governo, che ha esercitato la delega in maniera compiuta. Era stato dato questo principio di delega al Governo perché il nostro è un Paese nel quale ci sono circa 37.000 fattispecie di reato, in cui c'è l'obbligatorietà dell'azione penale il cui ingolfamento degli uffici giudiziari produce una lunghezza esasperante dei processi, che è l'esatto contrario della giustizia.

o no - sono scarse e limitate, quindi bisogna fare i conti e tutti i sistemi giuridici del mondo si fanno carico della limitatezza delle risorse, che impedisce di perseguire tutti i reati nello stesso modo, perché non è possibile.

aumentando i reati che possono essere non perseguiti per la particolare tenuità del fatto, affidando quindi al pubblico ministero o al giudice di valutare se la particolarità tenuità del fatto sconsiglia di perseguire un reato. Un altro strumento Un altro strumento è stata la depenalizzazione in concreto, perché se si leggono in tutte le riviste le osservazioni dei grandi luminari del diritto penale, tutti dicono che bisognerebbe depenalizzare.

introdurre nuovi reati. Qualunque questione sociale nel nostro Paese deve essere affrontata con un nuovo reato, perché è il modo più semplice per parlare all'opinione pubblica. Anche questa maggioranza non si sta sottraendo a questa tendenza, visto che - come diceva prima anche il collega Scalfarotto - ogni settimana siamo qui a discutere in Commissione di un nuovo reato. Quindi, di penalizzazione non si può parlare, perché nessuno è pronto ad assumersi la responsabilità di una depenalizzazione che sarebbe necessaria. Allora, cosa hanno fatto il Governo Draghi e la ministra Cartabia? Hanno cercato di fare quello che si può fare, e cioè una depenalizzazione in concreto: concreto: in alcune fattispecie, per alcuni reati, quando la persona offesa non ha l'interesse alla persecuzione del reo non si procede. Questa è la trasformazione di reati procedibili d'ufficio in reati procedibili a querela. Il problema che è stato posto, che in alcuni casi la persona offesa può essere indotta a non presentare querela, perché c'è un particolare condizionamento per il contesto in cui vive, è stato affrontato esattamente con questo disegno di legge, che noi condividiamo per questi aspetti, perché era necessario intervenire. Si tratta però di casi residuali, perché già oggi - lo voglio ricordare a tutti - anche per quei reati per i quali c'è stata la trasformazione in reati procedibili a querela, in caso di circostanze aggravanti si procede d'ufficio. Per esempio, le lesioni personali aggravate, la violenza privata o le minacce aggravate; aggravate; la minaccia grave, i delitti contro l'inviolabilità del domicilio, i delitti contro il patrimonio, l'appropriazione indebita, la truffa e la frode informatica sono tutti reati che, in presenza delle circostanze aggravanti, già oggi sono procedibili d'ufficio. nei quali sono coinvolti appartenenti ad associazioni criminali, di solito, quelli che oggi sono procedibili a querela e non più d'ufficio vanno insieme ai reati procedibili d'ufficio. veramente di casi residuali quelli nei quali è opportuno intervenire con questa norma, per fare in modo che non ci sia l'impunibilità. Ripeto: facciamo bene a intervenire, ma non enfatizziamo il problema, perché era già - secondo noi - abbastanza residuale.

che, in caso non sia presente la persona offesa dal reato in quel momento, quando c'è la flagranza di reato, si possa comunque procedere all'arresto, salvo la presentazione della querela entro le quarantott'ore successive. A noi - e non solo a noi peraltro, ma anche ad illustri studiosi di diritto penale - pare un corretto bilanciamento della necessità di evitare gli arresti indiscriminati - da un lato - e - dall'altro - anche i rischi di fuga o di inquinamento delle prove che altrimenti ci sarebbero. Quindi, tutto sommato, riteniamo che si tratti di una proposta di legge ragionevole che va a va a colmare alcuni vizi. C'entra gran poco con la riforma Cartabia che noi difendiamo, perché riteniamo che sia una riforma corretta che va nella giusta direzione. Per questo il Partito Democratico voterà a favore

le continue e qualificate sollecitazioni del Governo, da un lato, ma dall'altro il dibattito nell'Aula parlamentare e ancor prima quello in Commissione giustizia hanno confermato un dato pacifico, e cioè che le questioni legate alla giustizia sono tuttora un tema centrale per le forze parlamentari. Nel dispiegarsi di questa legislatura, che ha l'ambizione e la prospettiva di essere profondamente riformatrice, non va sottaciuto il dato che il tema della riforma della giustizia si ponga come una delle priorità per l'Italia. Questo perché, nel recente passato, abbiamo rischiato, sul tessuto connettivo della Nazione, un gravissimo vulnus. Abbiamo vissuto ore buie, abbiamo vissuto un interminabile conflitto tra politica e giustizia, che ha determinato veri e propri obbrobri giuridici,

ovvero il rischio di una deriva di una Repubblica giudiziaria fondata sull'azione penale, in cui la sovranità popolare fosse demandata alle procure della Repubblica che avessero titolo a esercitarla, talvolta in funzione della discrezionalità, quando non anche dell'orientamento politico. Tutto questo fortunatamente è oggi alle nostre spalle, perché il principio che ispira l'azione politica di Fratelli d'Italia è fare in modo che tutti gli interlocutori istituzionali - Governo, Parlamento, magistratura, avvocatura, accademia si ritrovino concordi, insieme, nel tentativo di raggiungere quel fine, invocato proprio l'altro giorno a Napoli dal Capo dello Stato, di avere finalmente un processo agile e moderno. agile e moderno. È in questa logica e in quest'ottica che si inserisce il disegno di legge che oggi andiamo a valutare e ragionevolmente ad approvare. La riforma Cartabia entrata in vigore partiva da un presupposto diverso rispetto all'ordinamento preesistente: ha aumentato a dismisura i reati procedibili a querela, rispetto a fattispecie che erano tipicamente procedibili d'ufficio, in funzione di un principio, quello della giustizia riparativa, che vedeva intorno alla persona offesa, intorno alla vittima del reato, non più un soggetto estraneo al protagonismo del processo, ma che ne faceva in qualche modo il cardine centrale. Il problema - alcuni problemi erano effettivamente addirittura preesistenti alla riforma Cartabia - è che, quando la riforma ha agito sul catalogo dei reati, ha finito col non interessarsi di taluni che richiedevano correttamente modifica e ne ha inseriti tali altri che invece hanno generato un fortissimo allarme sociale, perché avrebbero determinato vere e proprie forme di impunità. a prima firma del ministro Nordio interviene con grande equilibrio ed efficacia nel tentativo di fare in modo che ogni riforma da quella del singolo reato a quelle di sistema, fino a quelle di rilevanza costituzionale, separazione delle carriere, discrezionalità o obbligatorietà dell'azione penale, consacrazione dei principi del giusto processo - debba essere sempre declinata in funzione di due esigenze: tutela dei diritti del cittadino La riforma proposta dal ministro Nordio agisce chirurgicamente su alcune fattispecie laddove determinati contesti ad alto tasso di criminalità organizzata potevano in qualche modo condizionare la fruizione dell'azione penale attraverso l'istanza della querela di parte. Si tratta di un disegno di legge assolutamente chirurgico: sono solo quattro articoli, di cui peraltro uno relativo all'invarianza finanziaria, contenenti rispettivamente modifica al codice penale, modifica al codice antimafia, modifica al codice di procedura penale. con relazione agli articoli 270-*bis* e 416-*bis* si procede d'ufficio sempre - lo sottolineo - ogni qualvolta sia contestata l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ripeto: Articolo 2, modifica al codice antimafia: anche il delitto di lesioni personali deve essere sempre perseguibile d'ufficio ogni qualvolta sia commesso da soggetto sottoposto a misure di prevenzione e peraltro nell'arco di tre anni dal momento dell'esecuzione della misura. Articolo 3, modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale: consentire l'arresto obbligatorio in flagranza anche in assenza di querela, quando la persona offesa non sia immediatamente reperibile; più altre norme di coordinamento con il rito direttissimo e il rito direttissimo monocratico. È questo il percorso corretto: andare sempre a bilanciare le necessità di deflazione del carico giudiziario e di celerità dei processi con il primario dovere di tutelare la pubblica sicurezza. Uno Stato non può e non deve mai opporre la resa, la rinuncia, l'ignavia, la stasi, l'abdicazione rispetto allo specifico dovere di proteggere la collettività. E, quando parliamo di contesti mafiosi o di contesti terroristici; quando parliamo di sovraesposizione delle persone offese o dei cittadini e dei rischi di ritorsione; quando parliamo di clima di assoggettamento e di omertà legati alle associazioni criminali, noi abbiamo il vincolo profondo di proteggere i cittadini. E allora non c'è dubbio che la riforma vada coerentemente e coraggiosamente in questa direzione che dobbiamo conseguire non sono soltanto quelli della deflazione, a cui sono inevitabilmente connessi i fondi del Piano nazionale di ripresa Il tema è che proprio noi di Fratelli d'Italia, che siamo stati i più critici in passato rispetto a determinati orientamenti della riforma Cartabia, oggi la difendiamo per due ordini di ragioni: in primo va nella giusta direzione, quella di consentire finalmente allo Stato di esercitare fino in fondo la pretesa punitiva, andando a operare una scelta politica sulla procedibilità a querela; e poi soprattutto perché noi difendiamo la valenza degli accordi internazionali. E questo non perché gli accordi internazionali ci garantiscono, in funzione degli obiettivi, il diritto ad acquisire i fondi del Piano nazionale ma perché, attraverso il rispetto degli accordi internazionali, un Paese difende la propria credibilità. È questo ciò che vogliamo fare oggi. Allora - e con questo concludo sono finiti i tempi degli scribi e dei farisei, che oggi contestano la riforma astenendosi, quando fino a ieri hanno votato la legge delega in funzione della quale questa riforma questa riforma è stata approvata. *(Applausi)*. E si tratta di sepolcri imbiancati, che oggi gridano soltanto la loro ipocrisia. Oggi, Presidente, è il tempo della serietà e della responsabilità. Quindi, insieme al voto convintamente favorevole di Fratelli d'Italia, deve giungere un plauso al Governo, perché, in termini estremamente snelli, lineari sobri, è riuscito a sanare dei *vulnus* e soprattutto ha dato il senso della continuità a una lotta senza frontiere e senza tregua al terrorismo, alla criminalità organizzata e alle mafie di ogni dove e di ogni livello; un cancro invasivo e terribile che abbiamo tutti il dovere di combattere ed estirpare.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno della seduta. Passiamo pertanto alla discussione del disegno di legge n. 586,

Il 3 maggio scorso l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento. Pertanto la discussione sarà limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti e ordini del giorno, salve le dichiarazioni di voto finale. Il relatore, senatore Zanettin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. poc'anzi richiamato, di iniziativa dei senatori Romeo e Stefani, approvato in sede referente dalla Commissione giustizia, si propone di contrastare le truffe nei confronti delle persone anziane, fenomeno Il provvedimento - è opportuno ricordarlo - nella sua formulazione originaria era la riproposizione dell'Atto Senato 980, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura nel corso della passata legislatura. all'*iter* del disegno di legge, lei, signor Presidente, ha ricordato che, nella seduta del 3 maggio scorso, l'Assemblea del Senato ne aveva approvato, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, la procedura d'urgenza. Il provvedimento, inizialmente assegnato alla Commissione giustizia in sede redigente, a seguito della richiesta di un quinto dei componenti della stessa Commissione, è stato peraltro riassegnato alla stessa Commissione in sede referente. Nel merito, il disegno di legge si compone di un solo articolo, il quale apporta modifiche all'articolo 643 del codice penale, che riguarda la circonvenzione di incapace. Com'è noto, l'articolo 643 del codice penale, rubricato «Circonvenzione di persone incapaci», nella sua formulazione vigente punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque che, «per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso». L'articolo 1 del disegno di legge, nel suo testo originario, aggiungeva un ulteriore comma all'articolo 643, ai sensi del quale veniva punito con la stessa reclusione, da due a sei anni, e con la multa esattamente identica, da 206 a 2.065 euro, chiunque, al fine di procurare a sé o altri un profitto, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età all'età della persona, la induceva a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altro dannoso. della discussione, ha avuto modo di audire valenti giuristi, i quali hanno fatto emergere tutta una serie di criticità, alla luce della quale la Commissione ha ritenuto di apportare alcune modifiche all'articolo 1. 1. In primo luogo, si è intervenuti sulla collocazione sistematica della nuova norma, inserendola non più in un comma autonomo, bensì nell'ambito del primo comma dell'articolo 643 del codice penale. Ancora, sul piano della descrizione della condotta, sempre seguendo l'illuminato parere di valenti giuristi, si è ritenuto di riformulare, prevedendo che si configura il reato di circonvenzione di incapace anche nel caso in cui l'induzione della persona a compiere un atto dannoso, per lei o per altri, avvenga abusando delle condizioni di vulnerabilità, anche dovute all'età avanzata. è l'inciso che abbiamo apportato. La disposizione - è appena il caso di segnalarlo - riprende una formulazione già nota del codice penale. A ben vedere, infatti, l'articolo 61 del codice penale, sulle aggravanti, qualifica come aggravante comune l'avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Nel corso dell'esame in sede referente è stato invece soppresso l'articolo 2 dell'originario disegno di legge, sulla base di un emendamento identico del relatore e della senatrice Lopreiato, il quale interveniva sull'articolo 165 del codice penale, prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di truffa e di circonvenzione di incapace, la sospensione condizionale della pena per il reo fosse subordinata al risarcimento integrale della parte offesa. Questo perché, signor Presidente, è stata rilevata una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri reati, sempre contro il patrimonio, che però hanno una maggiore offensività e una maggiore pericolosità sociale. Mi viene in mente, Premesso che la mancata concessione della sospensione condizionale oggi consente comunque l'accesso al sistema delle pene sostitutive, la Commissione ha ritenuto che la previsione di un obbligo per il giudice di subordinare la concessione del beneficio all'effettivo risarcimento del danno, limitatamente ad alcune fattispecie di reato e non per altre della della stessa natura, potesse determinare una irragionevole disparità di trattamento, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione. La Commissione ha inoltre ritenuto che, in questi casi, fosse comunque più opportuno rimettere la decisione alla valutazione in concreto del giudice, in grado di poter apprezzare, caso per caso,

anche dovute all'età», si intende che quelle condizioni di vulnerabilità potrebbero riguardare anche altre persone che non siano anziane. Io ho proposto l'emendamento perché, se da un lato abbiamo certamente la necessità di tutelare gli anziani, dall'altro abbiamo anche la necessità di tutelare la certezza dei rapporti giuridici.

penso sia pericoloso. Preferirei che questo «anche» non ci fosse e che ci limitassimo alle condizioni di vulnerabilità dovute all'età, non solo avanzata, ma direi, al posto di «avanzata», «senile». questo aspetto perché dovremmo avere un'attenzione nella scrittura delle nostre norme. C'è una differenza tra l'età avanzata e l'età senile, e basta aprire il vocabolario: «avanzata» vuol dire che è avanti, ma avanti è un concetto molto ampio, relativo, soggettivo; invece l'età senile è un'età che ha a che fare con la senescenza della persona. Andiamo quindi a individuare la fattispecie del reato in modo più chiaro, aggiungendo alla situazione del minore, già prevista dalla legge, anche quella della persona - non anche, ma soltanto - che, data la propria età senile, si sia trovata in condizioni di vulnerabilità e, quindi, nella condizione di essere circuita. Mi pare che così chiariremmo meglio la portata della norma.

politiche serie di sostegno alle situazioni di fragilità che possono essere causate anche dall'età avanzata o comunque sicuramente in presenza di una situazione di fragilità. Il tema è il la circonvenzione di incapace è un reato da questo punto di vista affascinante perché sul tema dell'incapacità si dibatte molto. C'è ormai molta giurisprudenza ed è interpretazione pacifica che non è un'incapacità psichica psichica certificata, non è necessario, essendo sufficiente una situazione comunque di fragilità dovuta alle condizioni particolari di una persona o a una situazione di emotività che causa. È un problema di natura eminentemente sociale in una società che cambia. Siamo quindi nuovamente di fronte a un'iniziativa della maggioranza che ai problemi sociali risponde con norme penali. Questo invece è il classico terreno. Quando si parla di famiglia e si evoca la famiglia, cosa dobbiamo fare noi in una società che è cambiata e dove non ci sono più quelle reti familiari allargate che proteggevano gli anziani da - per così dire -incursioni? Noi dobbiamo creare delle altre reti; dobbiamo incoraggiare una rete di sostegno sociale costituita da parecchi attori da parecchi attori e interventi. Dobbiamo avere chiaro che il tema è la solitudine degli anziani, e non solo degli anziani. Dobbiamo farci carico della fragilità.

tutte le volte che gli interventi sono non dico conseguenti, ma esattamente nel senso contrario. Le esperienze non mancano su questo terreno. Ci sono Comuni e amministrazioni che hanno fatto campagne di informazione, hanno dato sostegno ad associazioni di volontariato e quant'altro, facendosi

ben poco. Noi vogliamo farci carico di queste fragilità; vogliamo creare una rete di sostegno affettiva e sociale; vogliamo dire che siamo consapevoli che la società è cambiata, ma non stiamo a guardare. Noi non proporremo a un anziano solo di abbracciare e di riscaldarsi con questa modifica legislativa. Noi vogliamo mettere delle persone fisiche a fianco di tali persone. Noi vogliamo davvero che questa

provvedimenti giustissimi come questo, ma che attengono in qualche modo a torti più gravi degli altri: penso ad abusi ai minori, alle persone con disabilità, ai cosiddetti anziani. Il mondo degli anziani è molto numeroso, per fortuna, e riguarda circa 14

in questa strana società dei *social*, che un pochino ci offende tutti anche se ci arricchisce di una nuova possibilità di comunicazione o perlomeno di parziale comunicazione,

di torti e di diritti speciali. Non è così: siamo tutti persone. Sembra banale ma lo dico anche per esperienza personale: sentirmi persona ci ho messo un po' di fatica perché, nonostante tutto, si deve dimostrare sempre qualcosa in più, una competenza in più, più volontà, essere più simpatici (cosa molto faticosa). E questa è violenza. Quante volte mi sono sentito dire: è disabile, ma anche onesto e ci mancherebbe altro. Come se certe qualità positive fossero giuste per le cosiddette persone normali, ma indispensabili per chi ha una disabilità, altrimenti: ci mancherebbe altro. Questo automatismo di competenze positive obbligatorie per chi mostra una qualche diversità io lo considero qualcosa di molto violento. Quanto agli anziani, di una razza a parte. Sono persone che per fortuna vivono di più; è una qualità positiva e lo dice chi, festeggiando quest'anno

E la voglio difendere per me e per chi non ha voce in capitolo. Lo dico sempre: quanti medici consigliano il fine vita a persone cosiddette imperfette, che invece sono portatrici di tanta gioia per se stesse e per gli altri? Detto ciò, considero l'attuale provvedimento ottimo, non solo perché giustamente punisce di più - e punire qualche volta è un deterrente indispensabile - ma perché ci permette anche in quest'Aula

perché, accanto ai danni che producono sulle persone anziane, ci vedo anche una mancanza di rispetto

la vita così preziosa di queste persone. Purtroppo - scusate il giro di parole - troppo spesso,

che riducono la memoria, la capacità critica, la capacità di reagire, non solo a livello motorio, ma soprattutto mentale. Vi è tuttavia qualcosa di peggio:

che si mascherano da esattori o che riceve belle fanciulle per avere chissà quali promesse, comprende di aver subito un reato anche un po' sciocco, si vergogna, non denuncia, perché più si cresce in età e anche nei pregiudizi delle persone cosiddette giovani, più si teme il giudizio delle persone, quindi si preferisce soffrire in silenzio piuttosto che chiedere qualche risarcimento. la psicologia di tutti, ma anche di queste persone tra cui ci sono anch'io, capiamo poco il valore di questo provvedimento, che sicuramente aumenta le sanzioni, ma ci permette di discutere su uno stato che dovrebbe essere positivo, quasi sacro, come tutte le fasi della nostra vita, ma che purtroppo spesso viene ridicolizzato. Accomunandomi

dirà, considerando in maniera estremamente positiva il disegno di legge in esame, credo che esista veramente qualcosa che non può essere sanzionato, ma che ci dovrà far riflettere a lungo: il vero reato che produce questi reati - e mi scuso ancora del giro di parole - è la solitudine.

per quanto possibile, anche la cultura dell'isolamento delle persone anziane, considerate una specie di categoria a sé, a sé, qualsiasi azione faremo sarà parziale. Io voglio che gli anziani vivano insieme agli altri in una realtà comunitaria, ci mancherebbe altro, ma prima di tutto che non vengano ristretti nella gabbia, nel carcere del pregiudizio che li obbliga a essere vissuti come persone da accudire e non come persone che in ogni caso manifestano una ricchezza

Presidente, sarò brevissima, anche perché sono già intervenuta in sede di discussione generale sul tema della tutela dei nostri anziani, che sono la nostra storia, ci trovi, per una volta, tutti d'accordo. Dichiaro quindi il voto favorevole dell'Alleanza Verdi e Sinistra al provvedimento in discussione. Si tratta di un disegno di legge già approvato nella scorsa legislatura, che interviene a modificare una norma penale finora non sufficientemente efficace sulla repressione di condotte quali truffe e raggiri particolarmente odiosi, perché commessi ai danni di soggetti fragili quali gli anziani. Il giudizio favorevole è anche frutto dei lavori fatti in Commissione e delle lievi modifiche al testo derivanti dai suggerimenti degli esperti auditi. Speriamo quindi di contribuire, con questo intervento, a rendere realmente efficace la risposta dello Stato a questa particolare tipologia di reato. Ad ogni modo, non vi è dubbio che occorresse intervenire di fronte alle frequenti notizie di truffe ai danni di persone anziane che, anche in ragione dell'attuale conformazione della società, spesso vivono da soli o comunque trascorrono gran parte delle loro giornate in solitudine. Vivono quindi una particolare condizione di fragilità dovuta all'età avanzata e a volte acuita da patologie di varia tipologia. L'abbiamo già detto: quelle riportate dalle cronache sono truffe i cui colpevoli si fingono operatori delle società di fornitura di luce, di gas e di acqua o addirittura delle Forze dell'ordine, che con scuse tutto sommato plausibili entrano nelle case di persone spesso sole e vulnerabili, le inducono a farsi consegnare soldi o beni di valore e le lasciano poi smarrite e confuse. Questi fatti hanno spesso sugli anziani un impatto emotivo che va ben al di là della truffa in sé. Non vi è alcun dubbio, infatti, che la vulnerabilità specifica che caratterizza l'anziano lo espone di fatto in maniera particolare al rischio di rimanere vittima di suggestioni, pressioni ambientali, influenze esterne, in altre parole a quell'attività di induzione a compiere atti giuridici di per sé dannosi che costituisce già uno degli elementi fondanti del reato di circonvenzione. Possiamo quindi ritenere che l'introduzione di una norma specifica dedicata al requisito dell'età avanzata sia una sorta di *alert* particolare, una lampadina che accendiamo e che, aggiungendo di fatto poco alla norma esistente, richiama l'attenzione del giudice su una particolare condizione anche in riferimento all'età della vittima. Pertanto, il provvedimento in discussione non rappresenta di certo una rivoluzione in ambito penale, quanto una sua più precisa definizione, andando a riempire in via legislativa una lacuna spesso già colmata dalle interpretazioni dei vari tribunali. È quindi con queste motivazioni che confermo il voto favorevole dell'Alleanza Verdi e Sinistra al provvedimento in discussione.

ma anche approfittare dell'occasione per puntualizzare, ancora una volta, alcune questioni che secondo me si stanno presentando con una certa frequenza in quest'Aula. e per suo tramite lo dico anche al Governo, che per tutta la durata della legislatura non cesserò di sventolare la bandiera rossa ed esprimere allarme circa la tendenza di questo Governo a mettere le mani continuamente nel diritto penale. è il secondo punto all'ordine del giorno ed è la seconda volta che mettiamo le mani nella sfera delle libertà dei cittadini.

tuttavia, non dobbiamo cadere nella tentazione di dare risposte all'allarme sociale che qualsiasi fenomeno provoca nel nostro Paese sempre con una norma penale. Voglio fare i miei complimenti ai colleghi del PD, i senatori Verini, Rossomando, Bazoli e Mirabelli, che hanno presentato l'ordine del giorno che da poco è stato accolto dal Governo, a cui

della loro solitudine, così come il tema della fragilità e del rischio che gli anziani corrono di essere vittime di raggiri proprio a causa di questa solitudine, non si risolvono soltanto con la norma penale. Bisogna essere accanto a loro, comunicare con loro e metterli in guardia dai rischi. Questo è il modo, secondo me, nel quale dovremmo provare a legiferare, altrimenti finiamo col mettere le mani sulle norme penali, sempre correndo rischi. Ho avuto modo di dirlo prima intervenendo sull'emendamento che avevo presentato e che non è stato approvato da quest'Aula, ma continuo a sottolineare che con quella parolina «anche», cioè dicendo che si può sollevare il

Allora, quel pezzo di carta, magari firmato in modo corretto, diventa più traballante, più instabile. La firma apposta su quel pezzo di carta diventa meno solenne e meno vincolante. Allora, capisco le buone intenzioni che ci sono dietro questa norma e le apprezzo così tanto da raccomandare al mio Gruppo di votare a favore della norma, però vi ricordo, cari

un fremito nella società, correre al codice penale. Guardiamo anche in modo più "olistico" a quali sono i problemi che ricorrono nella nostra società, che sono tantissimi. Se l'idea è sempre quella di tirare

sono veramente preoccupato di quale possa essere l'esito di questa legislatura. Una legislatura che era partita con tutta un'altra impostazione, perché - musica per le mie orecchie - il Ministro della giustizia si è presentato davanti a questo Parlamento sempre sostenendo il contrario dell'uso intensivo della norma penale. Ripeto, riconosciamo il bisogno di tutelare i nostri anziani e ammettiamo che, con una popolazione che invecchia sempre di più, il tema della

chi vive o ha vissuto con un anziano, chi lo frequenta o lo abbia frequentato, sa quanto, con l'aumentare della sua età, aumenti anche la sua vulnerabilità. Aumenta la sua debolezza fisica, spesso anche quella mentale, cioè, diventa più fragile. Nella società di oggi è certamente cambiato il ruolo sociale degli anziani, che non è più quello di una volta: quel ruolo, la conoscenza, la memoria, l'esperienza, che una volta erano considerati una testimonianza di saggezza all'interno delle famiglie, rischiano di venire meno quando l'anziano è lontano dai propri affetti. Purtroppo, in questo modo viene meno la rappresentanza di determinati valori ma anche quel prestigio sociale che si aveva una volta, di avere un saggio con i capelli bianchi in famiglia. Quando le persone avanti con gli anni vivono da sole diventano molto spesso più deboli e più vulnerabili. La politica deve quindi creare le condizioni per proteggerle, facendosi carico delle loro fragilità. L'allarme che riguarda gli anziani raggirati o truffati è, purtroppo, quotidiano. Spaventano i dati a loro riferiti. Se stiamo alle fredde statistiche che classificano anziani coloro che hanno più di sessantacinque vediamo che in Italia ce ne sono più di 14 milioni, e tra questi quattro milioni di ultraottantenni. Sembra un dato approssimativo quello di considerare anziano chi ha più di sessantacinque anni, quando conosciamo tante persone che hanno quell'età e sono ancora gagliarde. Sempre le statistiche del Ministero dell'interno ci dicono che il maggior numero di truffe nel 2022 è stato perpetrato proprio in danno di anziani uomini tra i sessantacinque Si tratta di quasi 26.000 reati a loro danno in un anno. Parliamo quindi di una media di 70 truffe o raggiri ogni giorno. Le insidie cui vanno incontro gli anziani sono soprattutto i reati al loro patrimonio, ma a quel punto, oltre al danno materiale, se ne aggiunge uno ulteriore: il danno psicologico infatti rimane, ed è di gran lunga più difficile da superare del danno economico. Proprio la trasformazione psicologica è quello che pesa di più su una persona fragile e avanti con gli anni, perché l'anziano subisce un'alterazione in un contesto sociale che dovrebbe proteggerlo, mentre, al contrario, lo colpisce di sorpresa. Ecco quindi che il problema non è tanto e solo quello del danno materiale: i soldi, i beni, i gioielli rubati, a cui si può quasi sempre porre rimedio. La cosa grave è il fatto che quella semplice sottrazione di un bene materiale fa sentire ancora più sola e fragile la vittima del raggiro. A quel punto ci si sente in balia di chiunque e non più in grado di condurre una vita sicura e dignitosa. In questi casi è stato rilevato che calano persino le difese immunitarie, si fanno sentire più pressanti le patologie esistenti e quasi non si riesce più a difendersi nemmeno da queste. Insomma, emergono una serie di problematiche ulteriori. Il senso più profondo della politica è proprio questo: aiutare i più deboli, chi non ce la fa, ponendo le condizioni affinché il contesto sociale in cui vivono sia loro più amico ed ospitale. Ecco perché questo disegno di legge, che contiene norme più cogenti sulla circonvenzione degli anziani, è assolutamente il benvenuto. Però va detto anche che la sola sanzione penale non basta e non sempre ottiene un effetto deterrente. La norma, ora migliorata e affinata, agisce solo dopo che il fatto è stato commesso in danno all'anziano. Noi crediamo che in questa sede il Governo debba prendere un impegno ulteriore nei confronti del Parlamento: quello di implementare una campagna per la sicurezza degli anziani, sia a livello nazionale che a livello locale. Ci sono tante informazioni che possono essere veicolate in modo che la vita dell'anziano possa essere più sicura. Auspichiamo pertanto che vengano promosse campagne via video e via radio che mettano in guardia dalle truffe e dai raggiri. Crediamo che un lavoro informativo ulteriore rispetto a quello che già svolge il Ministero dell'interno, per rendere più consapevoli gli anziani, possa essere fatto anche nei luoghi che questi frequentano quotidianamente. Penso, ad esempio, a campagne informative e distribuzione di volantini nei supermercati e nei negozi di prossimità, che rendano più consapevoli dei rischi, pur senza creare allarme. Bisogna cioè realizzare le condizioni affinché le fattispecie dei delitti che oggi andiamo meglio a specificare siano riferite a fatti che vedremo diminuire nel numero e nella pericolosità, grazie a un'appropriata e costante sensibilizzazione sul territorio. Intanto apprezziamo il disegno di legge che il Senato sta per approvare, a cui diamo il convinto voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

onorevoli colleghi e colleghe, il nostro sarà un voto di astensione sul disegno di legge di modifica del codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane, non perché non ne condividiamo l'intento, bensì perché non ne condividiamo il contenuto. Siamo a favore dell'offrire una maggiore tutela alle persone di una certa età, che in relazione a tale aspetto sono più vulnerabili al momento di compiere un atto dispositivo.

Siamo sicuri che la deficienza psichica di una persona, attualmente prevista dal primo comma dell'articolo 643 del codice penale, non normava già la condotta offensiva rivolta a soggetti di età avanzata e quindi maggiormente vulnerabili? O vogliamo pensare che questo disegno di legge vada a colmare una lacuna dell'ordinamento? Secondo noi, no. *(Applausi)*. Ma non solo secondo noi. Infatti la prevalente giurisprudenza ha precisato che, per l'esistenza di uno stato di deficienza psichica di una persona, non occorra una vera e propria malattia mentale, ma basti un'effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri. In tali circostanze, il giudice dovrà valutare se la condotta del soggetto agente sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi, secondo i criteri di normalità. Concludendo sul punto, già oggi in dottrina e giurisprudenza si è affermata la lettura del primo comma dell'articolo 643 del codice penale, che tiene in adeguata considerazione situazioni paragonabili a quella a cui si intende approntare tutela, poiché la deficienza psichica comprende tutte le ipotesi di minorata capacità intellettiva che possono rendere il soggetto facile preda dell'altrui opera di suggestione, non riconducibili all'infermità mentale, ma dipendenti da anomalie psichiche o situazioni fisiche. Situazioni fisiche quali la condizione di senilità di un soggetto. Ebbene sì, a legislazione vigente, tali condotte erano già previste. Vi è di più, però, e tale circostanza rende la maggioranza ancora più schizofrenica. Se da un lato, infatti, si interviene sul delitto di circonvenzione di anziani, dall'altro la conferma del regime di procedibilità a querela da parte della maggioranza per determinati reati crea un effetto paradossale. Per il vecchietto che subisce la violazione del proprio domicilio, che viene pestato a sangue e sequestrato, opererà il regime di procedibilità a querela. Quindi, si abbandona il vecchietto al proprio destino. Si lascia, infatti, alla capacità di un soggetto così indifeso la possibilità di ricorrere alla giustizia, in tal modo facendo sì che lo Stato si allontani inesorabilmente dal proteggere tale soggetto così vulnerabile. Un'ulteriore considerazione: abbiamo presentato pochi emendamenti, tutti nel merito, nessuno ostruzionistico e questo la maggioranza lo deve assolutamente riconoscere. Ne è stato approvato soltanto uno, soppressivo di un articolo. Su due articoli, la soppressione di un articolo mi sembra un buon risultato. Vuol dire che il 50 per cento del disegno di legge era sbagliato. Così come era sbagliata l'introduzione del delitto di *rave party*, la mancata modifica delle condizioni di procedibilità per alcuni gravi reati, con la restituzione del regime di ufficio, la mancata soppressione del concordato sui motivi in appello per alcuni gravi delitti, l'esclusione del patteggiamento tra le condizioni per ricadere all'interno della legge Severino, lo squilibrio del regime sanzionatorio per i percettori dell'assegno di inclusione sono alcune delle questioni che abbiamo messo al centro della discussione politica. Non ci avete ancora ascoltato, ma sono sicura che prima o poi lo farete. Ripeto che il nostro sarà un voto di astensione, perché vogliamo osservare come la giurisprudenza interpreta il novellato articolo 643 del codice penale e in quale rapporto si porrà quanto introdotto con il concetto di deficienza psichica, sperando

purtroppo, le notizie che riguardano episodi in cui sono state truffate persone anziane, coinvolte in raggiri

titoli più evidenti su casi di circonvenzione di anziano. Ravenna: raggira la parente novantenne e brucia 600.000 euro di patrimonio. Pinerolo: svuota i conti correnti di due anziane della parrocchia. tentano di rubare un anziano. Denunciati per circonvenzione di incapace. Riferisco solo i titoli, ovviamente non mi assumo le responsabilità di quello che viene esposto all'interno del giornale. Maltrattamenti aggravati, circonvenzione di incapace, violenze,

È facile, magari, che una persona si dica: «Il mondo è così complesso e può accadere che io non capisca». Può essere quindi che ci si trovi in queste situazioni. Sottolineiamo questo

qui entriamo nell'argomento oggi all'esame - la circonvenzione di persone incapaci. Sottolineo, per chi abbia dei dubbi, che attualmente la norma prevede la circonvenzione di persone incapaci.

abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona (...) la induce a compiere un atto».

parla proprio di circonvenzione di persone incapaci. C'è un *vulnus*, uno spazio che non è stato coperto dalla norma: sono quegli spazi grigi dove magari può trovarsi la persona

per chi è nato in un periodo in cui non si pensava minimamente che potessero esistere i cellulari), si trova oggi in un mondo estremamente complesso e di difficile comprensione. È per questa ragione che noi, come Gruppo Lega, abbiamo proposto il disegno il disegno di legge che porta la firma del nostro Capogruppo, l'Atto Senato 586. Esso nasce - lo sottolineo - da un dibattito che già si fece nel corso della precedente legislatura, perché la tematica è molto sentita. Poi i tempi della passata legislatura hanno impedito la trasformazione

di ascoltare le opinioni degli esperti sul tema. Ringrazio anche la presidente Bongiorno per aver saputo condurre un tema come questo che sembra facile, ma non è poi così scontato.

supportato da tutto un altro tipo di azione, come è stato proposto anche con il famoso ordine del giorno che avevamo discusso anche in Commissione giustizia, per far sì che queste persone siano supportate ed informate, grazie a strumenti che permettano di essere informati e di poter poter così difendersi non solo dalle truffe, che magari richiedono un impianto più complesso, ma anche da questi meccanismi molto diabolici che possono indurre le persone a compiere degli atti contro il proprio interesse e contro la propria volontà.

effettivamente ha assunto proporzioni sempre più preoccupanti. Credo che tutti quanti noi ne siamo in qualche modo testimoni per sentito dire o per parenti o per parenti che hanno subito tentativi di truffa telefonica o attraverso strumenti che ormai si stanno consolidando. Non c'è dubbio quindi che

per cercare di dare una risposta al contrasto di questi fenomeni, affrontandolo sotto il versante dell'intervento penale. Si interviene su una norma che già esiste, quella della circonvenzione di incapace,

facendo proprio, seppure attraverso una riformulazione, un nostro emendamento, ha messo mano a quel testo e ha fatto un lavoro accurato e condivisibile. Il testo iniziale infatti allargava per un verso, restringeva per un altro e creava qualche antinomia interna tra il primo e il secondo comma che viene introdotto. Il nuovo testo invece si limita a precisare meglio che quella fattispecie di circonvenzione di incapace si applica anche quando la persona che è indotta a fare qualcosa di dannoso per sé

ad evitare, come ci è stato segnalato da qualche audito, di immaginare una sorta di presunzione

e di truffe. Oggi siamo in una condizione molto diversa da tanti anni fa e quindi bisogna garantire anche alle persone anziane la piena libertà di volontà e di azione, quindi bisogna stare attenti. Tuttavia penso che questo miglioramento della norma sulla circonvenzione di incapace sia una scelta corretta: si precisa meglio la fattispecie e si chiarisce quanto, peraltro in parte, la giurisprudenza aveva già fatto, cioè che quella fattispecie si applica anche alle persone che sono vulnerabili in ragione dell'età. Siamo quindi favorevoli anche in ragione del fatto che è stata migliorata. Vorrei però che fosse chiaro a tutti se pensiamo, come in tutte le altre circostanze, di affrontare un fenomeno come questo solo sul piano della repressione penale, penso che rischiamo di fare un buco nell'acqua. Non è certamente esaustiva e risolutiva questa risposta, tanto per essere chiari, perché l'aumentare la pena da uno a due anni nel minimo e da cinque a sei anni nel massimo, per questo tipo di condotte, non penso che possa scoraggiare le persone che pongono in atto queste truffe. Va bene intervenire, va bene inasprire, va bene aumentare l'ampiezza della fattispecie, ma senza attribuire a questo intervento la capacità taumaturgica di risolvere il fenomeno: non è così e non possiamo girarci intorno. È un intervento opportuno, ma che non risolverà la questione. La questione si risolve - e noi avevamo presentato un emendamento in proposito (o si affronta in maniera forse più efficace e più adeguata) lavorando sulla prevenzione, cioè su tutto ciò che può aiutare a prevenire questi fenomeni: quindi con l'informazione alle persone anziane di stare attente a certi tipi di condotte e di telefonate, con una campagna pubblicitaria adeguata, con un supporto adeguato di sostegno alle persone sole. Questi sono gli strumenti più efficaci per tutelare le persone vulnerabili anche in ragione dell'età. Non pensiamo che, attraverso un inasprimento normativo di una sanzione penale, affrontiamo e risolviamo il problema. Va bene, facciamolo, siamo d'accordo, è stata fatta anche una norma tecnicamente corretta: ma certamente questo non risolverà il problema. Per tali ragioni, voteremo a favore, ma occorre fare molto di più.

onorevoli senatori, non vi nascondo che, ascoltando gli interventi dei colleghi in rappresentanza dei Gruppi che mi hanno preceduto, per un attimo mi sono illuso, perché ero convinto che probabilmente saremmo arrivati a votare questo provvedimento all'unanimità.

oggi all'attenzione dell'Assemblea, si propone di contrastare le truffe nei confronti delle persone deboli principalmente e - lo abbiamo aggiunto in Commissione,

Potremmo anche dire che un anziano potrebbe essere un diversamente giovane. Qual è la soglia che definisce che non si è più giovani e si rientra nella fascia degli anziani? Io ho apprezzato l'intervento del collega Guidi,

Si prevede addirittura che nel 2050 una persona su tre rientrerà in questi criteri, in ragione dei quali verrà considerata anziana.

cento rientra tra i casi di anzianità. L'Istat e la commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, istituita presso il Ministero della salute, hanno prodotto un rapporto sulle condizioni di fragilità e la domanda di assistenza sociale e sanitaria dei cittadini con almeno settantacinque anni. Quindi già passiamo dai sessantacinque I dati hanno evidenziato come su un campione di 6,9 milioni di ultrasettantacinquenni, oltre 2,7 milioni di individui presentavano gravi difficoltà motorie:

una questione sociale in questione penale. Non è così, perché probabilmente sfugge a qualche collega che non solo il Consiglio dei ministri

volte addirittura ad attuare le misure previste nel PNRR per le persone anziane non autosufficienti. Questo provvedimento è stato proposto direttamente dal presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, condiviso sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia dal Ministero

L'operazione ha portato alla luce una banda internazionale specializzata in truffe ed estorsioni ai danni di anziani e persone vulnerabili.

quando la critica è strumentale e addirittura proviene da chi oggi siede nei banchi dell'opposizione: da chi fino a ieri è stato non solo maggioranza, ma anche classe di Governo, quando la critica addirittura mette in evidenza delle spaccature all'interno dello stesso partito.

a un esempio fatto dal senatore Scarpinato in Commissione, che ripeto oggi: provate a immaginare quattro energumeni che entrano in casa di un anziano, lo malmenano e lo derubano. Aggiungo: provate a immaginare se in quel momento il vicino di casa chiama le Forze dell'ordine, che intervengono, colgono i malfattori in flagranza di reato e non li possono arrestare perché devono aspettare che l'anziano

le votazioni sul disegno di legge costituzionale riguardante lo sport, che richiedono un *quorum* qualificato, essendo la seconda votazione del Senato.

Colleghi, credo che questo Senato voglia ricordare il senatore Giorgio Bornacin, il 17 marzo scorso, dopo una lunga malattia, è venuto a mancare. Giorgio Bornacin era nato a Omegna, in Piemonte, ma da sempre viveva in Liguria; era genovese. Bornacin - lo ricordo - aderì giovanissimo al Movimento Sociale Italiano (alla Giovane Italia, per la verità, all'inizio), e al Fronte Universitario d'Azione Nazionale (FUAN) quando entrò in università. Agli inizi degli anni Ottanta divenne Capogruppo in Consiglio regionale regionale della Liguria per l'MSI e restò tale fino al 1996. In quegli anni fu il punto di riferimento del partito di Giorgio Almirante in Liguria. Nel 1994, quando quando c'è la svolta di Fiuggi, aderisce ad Alleanza Nazionale e, due anni dopo, diventa senatore; poi deputato nel 2001 e di nuovo senatore nel 2006 e nel 2008, quando nel frattempo

Ha lasciato in me un'impronta più grande perché era un mio grande amico, sostanzialmente quasi coetaneo, e con lui ho condiviso tante battaglie politiche. È sempre stato una persona garbata, ma inflessibile nei suoi convincimenti. Una persona che si è distinta per la sua coerenza, per il rispetto degli avversari e per la capacità di interpretare le proprie idee, adeguandole sempre al mutare dei tempi, ma conservandone la linearità. Con il senatore Gasparri - che parlerà dopo di me

politica attiva, la chiesa era stracolma di gente che non lo aveva dimenticato e che continua a serbarne il ricordo che merita. Ai suoi familiari, che ci hanno fatto sapere di seguirci attraverso il il video, e ai suoi amici, va il cordoglio mio personale e credo di tutto il Senato. Se lo ritenete, osserviamo un momento di silenzio in onore di Giorgio Bornacin.

Grazie, Presidente, per aver voluto questo momento di ricordo del senatore Bornacin. Il fluire delle generazioni e lo scorrere del tempo fanno sì che in quest'Aula forse solo alcuni abbiano avuto rapporti diretti, conoscenza, condivisione dell'attività parlamentare e, prima ancora, di quella politica. Alcuni di noi hanno avuto questo privilegio, lei per primo, come ha ricordato. Quindi è giusto che l'Aula del Senato, alcune settimane dopo la sua scomparsa, ne ricordi la figura. Le istituzioni

Nato in Piemonte, ha sempre vissuto e fatto politica in Liguria; ha sempre interpretato, dai lavoratori frontalieri ai temi della portualità e dei trasporti, un'azione politica

Voglio ricordare qui Giorgio Bornacin, in un'epoca in cui la selezione nella politica e i *social*, tanti mezzi più rapidi, determinano a volte un andare diverso della politica. Ma c'è anche una politica che nasce nella militanza, nell'impegno negli organismi universitari e nelle scuole, nel Consiglio regionale, dove Bornacin fu eletto e membro dal 1980 al 1996, fino a quando, secondo un percorso (una volta si faceva così), approdò in Parlamento. Ha condiviso con molti di noi tutti i passaggi di trasformazione della destra politica. Il padre, dirigente politico della destra, gli aveva indicato un orizzonte di valori che Giorgio Bornacin non ha mai tradito. Uomo sicuramente appassionato delle sue idee, ha fatto parte di uno schieramento politico: quindi era uomo di parte nel senso nobile e fiero della parola. Quando è venuto a mancare prematuramente, a causa di una serie di vicissitudini, di malattie e di affaticamento fisico precoce,

molto appassionato. Coloro che non solo in quest'Aula, ma a Genova e altrove, ci stanno ascoltando attraverso i mezzi che ci consentono di raggiungerli, apprezzeranno certamente questo ricordo da parte dell'Aula del Senato, così come di tutte le istituzioni politiche, tra cui la Regione Liguria e la Camera dei deputati, che lo aveva ricordato alcuni giorni fa.

libri e volumi dedicati alla storia della militanza della destra genovese e alle vicende di Ugo Venturini, una delle prime vittime degli anni di piombo. Venturini era un lavoratore che a Genova cadde nel 1970, durante un'aggressione a un comizio del Movimento Sociale Italiano. Giorgio, anche su queste vicende, come su tante altre di volontari italiani caduti all'estero, ha mantenuto un filo con le famiglie, in un'azione di rispetto dei valori nazionali che non ha mai abbandonato. Quindi concludo questo ricordo con commozione, perché per molti di noi Giorgio Bornacin ha rappresentato un pezzo di vita, un percorso

il lavoro e la figura di Giorgio Bornacin. Giorgio Bornacin ha svolto, come giustamente lei ha ricordato nel suo intervento, moltissimi ruoli dal punto di vista istituzionale. È stato, appunto, componente del Consiglio regionale della Liguria ed è stato per moltissimo tempo deputato e senatore. Io lo ricordo come avversario, perché è sempre stato schierato con idee e da una parte politica che era oggettivamente lontana dalla mia. Però, proprio da amministratrice della Regione Liguria, ho potuto apprezzare la sua lealtà, il suo senso delle istituzioni e soprattutto - ci tengo moltissimo a dirlo - la sua capacità reale di occuparsi dei problemi veri del suo territorio. Di Giorgio Bornacin ricordo le battaglie incredibili nei confronti dell'isolamento della Regione Liguria e la sua battaglia per le infrastrutture. Ricordo i suoi interventi in favore della realizzazione del terzo valico dei Giovi. Ricordo quella capacità, che solo i politici che vengono anche dal territorio in fondo hanno, di costruire relazioni e una volontà di sintesi anche con le parti politiche avverse. Questa lealtà istituzionale, questo amore nei confronti del territorio, questa grande passione ideale nei confronti della propria comunità sono il ricordo più bello e prezioso che porto con me: di una figura che è stata sicuramente lontana dalle mie posizioni politiche, ma mai un nemico, mai una figura con la quale avere delle polemiche sterili, perché al primo posto, per Giorgio Bornacin, c'era sempre l'interesse della Liguria e l'interesse del Paese. Per questa ragione ci piace ricordarlo oggi, perché veramente credo egli abbia, per una lunghissima fase della sua attività amministrativa e istituzionale, svolto un ruolo prezioso per tutta la comunità. Signor Presidente, di Giorgio Bonacin, ex parlamentare e consigliere regionale genovese, viene ricordato che il suo percorso politico è sempre stato ispirato dai propri ideali. Nonostante fosse un uomo di contrapposizione, anche gli avversari politici ne rispettavano la determinazione e l'onestà intellettuale. Ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso politico, il sincero cordoglio del Gruppo MoVimento 5 Stelle del Senato.

con affetto e sentimento, a prescindere dall'appartenenza politica. Come è stato detto in questa sede, egli era sicuramente un uomo di parte, riconosciuto come coerente rispetto ai suoi ideali e ai suoi valori, per cui ha speso una vita. È stato, però, un uomo politico estremamente rispettato da tutti, dagli avversari Grazie per quattro volte parlamentare della Repubblica e per moltissimi anni protagonista della vita amministrativa, anche se all'opposizione, della sua Regione, per la quale si è sempre battuto, com'è stato ricordato: dal tema dei portuali alle questioni legate alla sua comunità. Forse, però, il ricordo più bello, anche per la sua famiglia, cui esprimiamo il cordoglio come Gruppo Partito Democratico, è il ricordo di una persona sempre disponibile per la comunità: per la sua comunità cittadina, per i suoi amici, per la sua parrocchia. Una persona vicina al suo territorio e vicina alle istituzioni, che ha rappresentato per moltissimi anni.

identificato la politica di vecchio stampo, che, al di là delle differenze di vedute politiche, ha sempre visto il rispetto degli avversari politici. L'amore per la Liguria è quello che lo ha sempre contraddistinto nella sua attività politica.

mi ha convinto, insieme ad altri, a fare politica da giovane - che un giorno avrei avuto l'onore di commemorarlo nello stesso luogo in cui ha svolto parte della sua carriera parlamentare. Sono foto sbiadite, che ci riportano al Movimento Sociale degli anni Ottanta; altre, un po' meno sbiadite, ci riportano all'avventura in Alleanza Nazionale e poi, ancora, al PdL, come giustamente ha ricordato anche lei, signor Presidente, e come ha raccontato l'amico di Giorgio, Maurizio Gasparri.

fortemente avversari, esponenti dell'ex PC genovese, che hanno deciso di rendere omaggio a un uomo leale, che non si è mai scostato dalle sue posizioni, ma che le ha sempre sostenute lealmente e ha sempre combattuto per poterlo fare. Parliamo di un uomo che è nato in un certo tipo di destra, nel Movimento Negli anni Ottanta è stato il referente ligure di Giorgio Almirante; è stato anche il mio referente politico, prima in Regione e poi in Parlamento. È stato un uomo che, com'è stato già detto, adeguare le proprie idee al cambiamento dei tempi e ha accompagnato il lungo percorso della destra italiana, che dalla protesta è passata alla proposta, dalla proposta al confronto e dal confronto alla sua modifica genetica fino alla svolta di Fiuggi cui Giorgio aveva aderito con grande entusiasmo. Giorgio ci ha consegnato e ci consegna una destra moderna, profondamente cambiata ed evoluta nei tempi; devo dire che, se oggi Fratelli d'Italia è al Governo della Nazione, lo si deve anche a uomini come Giorgio, che hanno saputo interpretare la storia della destra, dal Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale e poi al PdL, fino alla nascita - anche se lui in Fratelli d'Italia non è mai entrato - dell'attuale destra di Governo. Sono certo che lassù, dove Giorgio sarà e dove avrà incontrato gli amici di tante battaglie aspre e dure e anche tanti avversari, sarà felice di averci permesso di essere qui in Parlamento a rappresentare quelle che sono state anche le sue idee. Ciao, Giorgio.

l'Istituto comprensivo «Dante Alighieri» di Leonforte, in provincia di Enna, paese che conosco anche di persona.

in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previe dichiarazioni di voto.

Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, esprimo anzitutto la mia soddisfazione perché ci troviamo qui per la seconda volta, a distanza di pochi mesi, in quest'Aula a dare definitivo "disco verde" all'approvazione di un provvedimento che, al termine dell'ultimo passaggio nell'altro ramo del Parlamento, conferirà finalmente rango costituzionale allo sport italiano, come già abbiamo fatto con animali e ambiente, riconoscendo il suo alto valore all'interno della nostra Carta costituzionale, richiamandosi a quella definizione di sport che il Consiglio europeo aveva già evocato sin dal lontano 1992. un passaggio - lo dico avendo avuto l'onore di essere stata Sottosegretario allo sport - non certo simbolico, ma anzi connotato dalla forte consapevolezza che questo Governo, e con esso l'intero Parlamento, si è assunto un impegno chiaro ed una responsabilità chiara: tributare a tutto il sistema sportivo italiano, ai dirigenti, ai praticanti e alle istituzioni che lo animano, il giusto riconoscimento per i valori e i meriti che sono stati capaci per usare una metafora sportiva - di sudarsi e guadagnarsi sul campo. Grazie anche a loro, al CONI e al suo energico presidente Malagò, è arrivato uno stimolo paziente e continuo, prontamente colto dal ministro Abodi e da una maggioranza in sintonia e attenta alle trasformazioni della società. Non dobbiamo però incappare nell'errore di considerare questa riforma della nostra Carta costituzionale, che introduce lo sport all'articolo 33, come un punto di arrivo. Essa è, al contrario, un punto di partenza, un primo passo a cui la nostra Repubblica deve impegnarsi a dare sostegno. Questo provvedimento si inserisce quindi nell'alveo di altre importanti riforme che questo Governo e questa maggioranza hanno intrapreso, dalla stabilizzazione dei docenti di educazione motoria nella scuola primaria, passando per alcune agevolazioni anche fiscali, come la prescrizione dell'esercizio fisico strutturato a soggetti con patologie croniche non trasmissibili, sino alla detraibilità delle spese per l'attività fisica privata a scopo di prevenzione. L'attività sportiva entra quindi nella nostra Carta costituzionale con la stessa dignità con cui da sempre aiuta la nostra società a diffondere i valori di solidarietà, lealtà, sacrificio, rispetto delle regole, *fair play* e rispetto della persona. Questa riforma ha poi il merito di occuparsi di un aspetto non proprio secondario delle nostre vite, quello della salute, del *buen vivir*, della *healthy care*, soprattutto se pensiamo a questi ultimi anni: anni di pandemia e di isolamento sociale; anni pesantissimi, che indubbiamente hanno avuto ripercussioni fortissime sull'educazione e sulla socialità dei nostri figli, dei nostri bambini e dei nostri giovani,

però consapevoli che deve corrispondere allo stesso modo un dovere da parte dello Stato nei confronti della società, quello di rendere lo sport accessibile a tutti, a prescindere dalle condizioni sociali ed economiche e dalla fascia d'età, prestando particolare attenzione al tema delle disabilità e - vorrei aggiungere - anche dei lavoratori dello sport, che hanno bisogno di ulteriori tutele, perché perché sono lavoratori a tutti gli effetti. In altre parole, vogliamo che il diritto allo sport diventi a tutti gli effetti universale, poiché lo sport rappresenta un minimo comune denominatore capace di abbattere muri e barriere, uno strumento forte per perseguire il progresso e lo sviluppo individuale prima di tutto. La stessa Carta olimpica, nell'elencare i principi fondamentali dell'olimpismo, ce lo insegna e sancisce che la pratica sportiva è un diritto dell'uomo e che a ciascuno dev'essere riconosciuta la possibilità di esercitarlo senza discriminazioni. Lo sport, praticato a livello tanto agonistico quanto dilettantistico, unisce e insegna ad affrontare il gioco di squadra, a perseguire il rispetto delle regole, a sopportare i sacrifici, a proporsi obiettivi, a gioire per le vittorie e ad accettare le sconfitte. Lo sport è educativo per tutta la società e dovrebbe essere molto d'esempio ai nostri giovani. Promuovere la pratica sportiva e l'attività motoria e tutelare scopi ed interessi deve rappresentare al tempo stesso un obiettivo politico di lungo periodo e l'impegno che vogliamo assumerci nei confronti di quanti attribuiscono allo sport sport importante rilievo nella formazione individuale e guardano ad esso quale veicolo per diffondere valori come l'uguaglianza, la lealtà, la parità di genere, il sacrificio e lo spirito di squadra: ciò nell'ottica di un approccio collaborativo e di sana competizione, a cominciare dalle buone pratiche nella scuola primaria, l'unica vera palestra per la salute psicofisica delle nuove generazioni. Non è che l'inizio, si diceva. A questa cornice costituzionale vogliamo aggiungere un contenuto chiaro e coerente, quali, ad esempio, il potenziamento dei progetti sugli studenti atleti e dei licei sportivi, il rafforzamento dell'offerta territoriale, l'introduzione nelle scuole di ogni ordine di materie che promuovano la cultura dello sport e non soltanto l'attività motoria, e così discorrendo. Il nostro Gruppo parlamentare Civici d'Italia-Noi Moderati (MAIE-UDC)-Coraggio Italia, e questo Governo con noi, ha chiaro il concetto che solo ricostruendo un rapporto sano, virtuoso, organico e strutturato con il mondo della scuola scuola si potrà dare, anche alla pratica sportiva, la giusta dignità che merita. È un lavoro certamente lungo, ma grazie a questa riforma sono maturate certamente una maggiore consapevolezza politica e una sensibilità riguardo alla sua fondamentale importanza. Siamo certi che, anche grazie al prezioso contributo dei comitati italiani olimpico e delle federazioni, dei gruppi sportivi militari, delle società sportive e dei loro allenatori e tecnici, il nostro sistema sportivo italiano potrà essere più forte e più competitivo e arrivare laddove sino ad oggi non è riuscito ad arrivare. Non dimentichiamoci però che il sistema sportivo italiano non è soltanto lo sport di vertice. Esso poggia quotidianamente sul sacrificio, sull'esperienza, sulla professionalità e sull'abnegazione di centinaia di migliaia di persone, di dirigenti, di presidenti di associazioni sportive, di volontari, di istruttori, di allenatori e di quel milione circa di lavoratori sportivi che, nonostante tutto e nonostante le difficoltà, si sostituiscono - per così dire - a un presidio dello Stato, tenendo aperti i centri sportivi nei quartieri più periferici e degradati dei nostri centri urbani, oppure animando le piccole palestre e le scuole dei nostri Comuni, allenando ed educando

Volendo usare un'altra metafora sportiva, sebbene il loro lavoro sia sempre stato lontano da quei riflettori da stadio, essi meritano una medaglia d'oro al valore e al coraggio, perché sono in grado di educare, crescere e migliorare le future generazioni dal punto di vista non solo del benessere psicofisico, ma appunto di quei valori intrinseci e fondanti di ogni società sana. Non dimentichiamoci altresì che quella sportiva è un'attività di fondamentale importanza per l'economia del nostro Paese, un settore in grado di generare circa 100 miliardi di euro l'anno e ad alto moltiplicatore sociale, se pensiamo che perseguire uno stile di vita sano diminuisce il rischio di patologia in età avanzata, e ciò favorisce quindi una maggior razionalizzazione della spesa pubblica sanitaria con evidenti ricadute positive sulle casse dello Stato. Signor Presidente, mi lasci poi dire che questa riforma non avrebbe mai visto la luce dopo tutti questi anni di attesa, senza la caparbietà e l'iniziativa di alcuni colleghi senatori di maggioranza, come pure del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché, da donna coerente qual è (com'è sempre stata, continuando a dimostrarlo a tutt'oggi ed essendo ripagata dagli elettori), ha manifestato sempre grande attenzione e sensibilità al tema dello sport, sia dai banchi dell'opposizione sia oggi alla guida di questo Governo. Non era certamente una cosa scontata: infatti, dopo anni in cui le speranze e con esse anche le risorse delle politiche pubbliche destinate allo sport sono state ridotte ridotte al lumicino, questo Governo guidato da Giorgia Meloni ha eroicamente avviato un percorso di ricostruzione di un'armonia istituzionale tra il mondo politico e quello sportivo. alla conclusione, signor Presidente. Inclusione, integrazione, valore sociale, prevenzione, sicurezza, economia: lo sport è capace di sintetizzare in una sola parola tutti questi termini. La sua cristallizzazione nella Carta fondamentale dei valori della nostra Repubblica non potrà che riconoscergli, quindi, un valore universale. Oggi voltiamo finalmente pagina e confermiamo di voler elevare lo sport quale diritto imprescindibile, fattore di aggregazione e formidabile veicolo di inclusione sociale. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con

Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, la modifica dell'articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva prevede che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico

Da ultimo, nella seduta dell'Assemblea dello scorso 29 novembre, è stata approvata la richiesta di procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, che riguarda il disegno di legge n. 13. Sappiamo bene che lo sport in tutte le sue forme rappresenta un importante strumento formativo, di integrazione sociale e di diffusione di valori universali positivi, e un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale. Per tutelare il diritto all'accesso di tutti senza distinzione allo sport, già desumibile dall'articolo 2 della Carta costituzionale, è però necessario mettere in campo risorse e modalità di sostegno anche agli enti locali e investire ancora di più da questo punto di vista nell'ambito dell'istruzione. Infatti, l'impossibilità di praticare lo sport colpisce in Italia circa un minore su cinque, che, tra i sei e i diciassette anni, non pratica sport non pratica sport e il 15 per cento svolge solo un'attività fisica. Questo però è il frutto di una povertà economica diventata ormai vera e propria emergenza; non è il frutto di riforme, ma di mancati investimenti, che purtroppo riguardano soprattutto la scuola. Alla povertà economica si intrecciano irrimediabilmente la povertà educativa, investimenti in istruzione insufficienti, edifici poco sicuri e tassi di abbandono scolastico altissimi. Vorrei fare però una precisazione. Se si vuole ribadire l'importanza dello sport, non c'è bisogno di rendere farraginosa e stratificata la nostra Carta costituzionale, che le nostre madri e i nostri padri costituenti ci hanno lasciato in eredità, ma è necessario ampliare i servizi gratuiti per accedere alle attività sportive e curare gli spazi verdi dei centri e delle periferie delle nostre città, per consentire a tutti di svolgere attività fisica all'aperto, ancor di più oggi, dato che l'isolamento prolungato dovuto alla pandemia ha accresciuto in maniera preoccupante tendenze già in essere tra i più giovani: isolamento, disagio emotivo, sregolatezza, ansia, depressione, difficoltà di concentrazione, disturbi alimentari, insonnia, sfiducia in sé stessi e nel futuro, dipendenze dai *social network* e dai videogiochi, oltre che da alcol e droghe, nonché ritiro sociale, aggressività e autolesionismo.

sullo sport in genere la cifra dovrebbe essere di 700 milioni di euro. Bisogna però vigilare che, all'interno dei bandi che si faranno, venga ripartita la quota almeno del 40 per cento al Sud prevista dalla normativa vigente è su questo che dobbiamo concentrarci anche per far sì che quella presente possa diventare un'importante occasione. Qualche mese fa, nella scorsa legislatura, è stata promulgata la riforma costituzionale che modificava gli articoli 9 e 41 della Costituzione, inserendo tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, con un patto intergenerazionale. Come lei e i suoi colleghi comprenderete, stiamo parlando di una questione che riguarda il futuro dell'umanità e delle specie viventi, vista l'emergenza climatica e ambientale. Faccio questo riferimento perché, nella discussione che si è avviata su quella riforma molti costituzionalisti hanno detto che, nonostante fossero d'accordo sull'inserimento della tutela ambientale, avrebbe potuto esserci il rischio di favorire in questo modo interventi *spot* sulla prima parte della Costituzione. Ebbene, dopo poco tempo si è pensato di introdurre questa ulteriore riforma. Ciò che dico riguarda non già il valore fondamentale dello sport, bensì il rischio molto forte di iniziare un periodo di microinterventi puntuali sulla Costituzione in cui ognuno si attiene alla questione che più gli sta a cuore. Penso che andrà fatta una riflessione sulla necessità di evitare che si possa intervenire in questo modo sulla prima parte della Costituzione, ossia su quella più progettuale e programmatica e non sui suoi principi fondamentali. Credo che dobbiamo fare questa riflessione in modo approfondito per evitare che si possa dar vita a una stagione di micromodifiche costituzionali in cui ogni parte, ogni parte, partito o Gruppo che lo voglia possa portare all'attenzione temi dei quali si ritiene necessario un riconoscimento costituzionale. Per questi motivi, Alleanza Verdi e Sinistra ci asterremo, fermo restando che davanti alla Costituzione ognuno ha la libertà di esprimersi come ritiene,

è molto importante che questo comma che andiamo a inserire nella Costituzione vada a integrare l'articolo 33, cioè quello che prevede la possibilità per la Repubblica di garantire l'istruzione dei nostri concittadini, soprattutto dei giovani, con riferimento in particolare all'arte e alle scienze e quindi pone sullo stesso piano per la vita dell'uomo di oggi e soprattutto degli uomini e delle donne di domani

misura minore nell'ambito scolastico e gli insegnanti di educazione fisica - non lo scopriamo oggi - si sentivano un po' l'ultima ruota del carro nel collegio Adesso non lo saranno più, perché svolgono un'attività che la Costituzione individua come fondamentale. Questo secondo me è molto importante e ovviamente dovrà avere seguito con una riorganizzazione dell'attività scolastica, questo è già un buon punto di partenza. Non dimentichiamoci che c'è un problema storico in Italia di convivenza negli istituti scolastici e nelle palestre tra l'attività scolastica vera e propria e quella delle società sportive, che spesso è un rapporto che porta ad avere difficoltà e a creare contrasti. Ebbene, con questo passaggio della Costituzione si spera che questi contrasti potranno essere limitati, perché le società sportive hanno il pieno diritto di fruire di impianti e strutture pubbliche, al pari dell'attività scolastica vera e propria. Mi permetta, signor Ministro, di sottolineare che la formulazione stessa di questo comma è

Lo sport ha la possibilità di tenere i giovani uniti, di metterli insieme e di inculcare in loro valori positivi: etica, rispetto delle regole, uguaglianza, lealtà e senso della meritocrazia tutte cose che altrimenti rischiano di non essere oggetto dell'educazione nell'età giovanile, che è quella che poi determina la personalità di ciascuno. Vi è poi il «valore sociale» dello sport: viviamo nella società dell'isolamento da *smartphone*, in cui cui è possibile che ciascuno viva per conto proprio quasi tutte le ore della vita da sveglio, perché quando dorme vive da solo comunque. Allora, nella società di questo autoisolamento, lo sport costringe le persone a stare insieme e fare cose insieme, favorendo soprattutto nei giovani, ma non solo, virtù come la pazienza e la capacità di accettare l'altro e di concentrarsi, cosa che manca molto oggi nelle scuole. Nello sport non esiste, al contrario dei videogiochi, il *game over*; si riparte sempre un'altra volta, quindi chi perde oggi può sempre sperare di vincere domani. Poi si parla della «promozione del benessere psicofisico» e quindi della prevenzione di malattie, sia del corpo sia della psiche, che sono foriere di malessere sia per i singoli individui, sia per coloro che vivono loro vicino. Soprattutto, è un modo per prevenire costi pubblici e sociali. «in tutte le sue forme»: questo è un passaggio fondamentale, perché si tratta di sottolineare che lo sport non è soltanto attività agonistica degli atleti o delle squadre di vertice, ma è tale a tutti i livelli, agonistici o amatoriali. La mano pubblica in tutte le sue articolazioni, in particolare nei Comuni, è in questo modo non solo legittimata, ma anche indotta ad investire di più e a destinare più risorse per la realizzazione e il mantenimento di impianti sportivi. È una scelta felice per tanti aspetti, ma soprattutto consente

l'avremmo già potuta approvare nella scorsa legislatura. Senza fare polemiche, voglio solo ricordare che quel Governo è caduto prima, altrimenti avremmo già portato a casa questa modifica costituzionale.

aggiunto quel comma all'interno dell'articolo 33 della Costituzione, relativo al diritto all'istruzione, ma anche accanto all'articolo 32 della Costituzione, relativo al diritto alla salute. Le due cose stanno esattamente insieme ed è un binomio perfetto: com'è stato detto da tutti i colleghi che mi hanno preceduta, salute e sport e sport è un binomio fondamentale e il pilastro stesso per costruire una vera riforma del *welfare*. Vogliamo Vogliamo infatti riconoscere pienamente - ecco perché andiamo a modificare la nostra straordinaria Costituzione - che anche l'attività sportiva possa diventare un diritto universale, di tutti e per tutti. Ciò non è ancora scontato, purtroppo, nella nostra società e il Covid ha anzi contribuito ad aumentare le diseguaglianze sociali, culturali,

soprattutto tra i bambini più piccoli. Ecco perché oggi questa modifica costituzionale ci consente finalmente di arrivare a un sistema di *welfare* completo, che oggi ancora non c'è, in cui anche i fondi

com'è nei pensieri e nelle azioni del ministro Abodi. È una riforma importante, che si unisce a quelle dello sport, che entrerà in vigore il 1° luglio.

è il riconoscimento di un diritto universale di inclusione sociale e di integrazione, fondamentale nella scuola e nella prevenzione, ma aggiungo anche nel contrasto alle dipendenze. a quei Paesi che - soprattutto se guardiamo al Nord Europa - hanno potuto abbattere del 50 per cento dipendenze dovute all'alcol o alla droga proprio attraverso l'attività sportiva.

sul riconoscimento dello sport come farmaco da prescrivere in ricetta medica. Si tratta di un provvedimento importante, che il ministro Schillaci, insieme al ministro Abodi, ha voluto ribadire come fondamentale anche nelle prossime scelte del Governo, e noi siamo contenti come parlamentari di aver contribuito a ciò, prevedendo anche detrazioni fiscali: se vogliamo aiutare le famiglie e i soggetti più deboli che oggi non si possono permettere di fare attività sportiva, anche questa misura va loro incontro, da questo Penso a detrazioni fiscali nel modello 730, come facciamo per i farmaci: attraverso questa modalità trasparente e chiara potremmo farlo anche per un abbonamento a una palestra, a una piscina o a qualunque attività sportiva. poi il grande tema del professionismo femminile, a cui teniamo moltissimo e per cui ci siamo battuti anche nella scorsa legislatura. Oggi il professionismo femminile è riconosciuto soltanto nel mondo del calcio: dobbiamo fare in modo che questo importante riconoscimento possa abbracciare tutti gli sport. confrontati molte volte - è importantissimo - così come sta già facendo all'interno della riforma dello sport - che ci sia una distinzione netta tra il mondo del professionismo e il mondo del dilettantismo. Sono ovviamente due modi e due modelli diversi, entrambi fondamentali; entrambi contribuiscono all'economia e all'aumento dell'occupazione. Penso soprattutto al lavoro sportivo, al riconoscimento di molte professioni che oggi, nel mondo sportivo, non sono ancora riconosciute.

permettetemi di parlare di un altro tassello che si è aggiunto: il riconoscimento dei laureati in scienze motorie nelle scuole. I fondi non sono ancora sufficienti. Qui mi appello al Governo affinché si possano assumere altri laureati in scienze motorie e affinché lo sport venga riconosciuto come materia scolastica a tutti gli effetti. Non possiamo lamentarci se l'Italia non ha i vivai ed è al primo posto solo quando vince

anche a livello di istruzione e di scuola. Il lavoro da fare da questo punto di vista è tantissimo. Noi ovviamente ci siamo, ci saremo e voteremo a favore di questa importante modifica costituzionale.

culturale e sportivo. Quanto potrebbe incidere sul PIL del nostro Paese? Più andiamo a sportivizzare le nostre comunità e i nostri Comuni,

dal Parlamento e ringraziando il ministro Abodi per la sua sensibilità e per le azioni che ha già messo in campo. questo disegno di legge costituzionale torna per la seconda deliberazione al Senato, con l'intento di valorizzare l'attività sportiva tra i principi della nostra Costituzione. una modifica all'articolo 33, aggiungendo un comma che recita: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva Lo sport e l'attività sportiva hanno assunto un'importanza fondamentale nella vita quotidiana di ogni essere umano, giovane e meno giovane.

di ordinamento sportivo. Oggi, finalmente, siamo vicini al traguardo di inserire nella nostra Costituzione il riferimento alla pratica sportiva. Forza Italia è assolutamente favorevole a questa modifica costituzionale, poiché ritiene che sia fondamentale conferire una dignità ancora più alta allo sport e a tutto ciò che l'attività sportiva rappresenta. perché lo sport è benessere, perché contribuisce, in modo fondamentale e spesso insostituibile, al benessere fisico e psicofisico delle persone. Lo sport è fondamentale per è fondamentale per il benessere psicofisico delle persone con disabilità. Ho visto persone tornare a sorridere, tornare ad aver voglia di vivere, capire che si può diventare campioni anche se si hanno problemi fisici. Lo sport è anche salute e, per questo, contribuisce a razionalizzare e a far diminuire la spesa sanitaria, riducendo il ricorso alle strutture sanitarie. L'attività sportiva è utile nella cura di alcune malattie ed è fondamentale nell'aiuto di alcune disabilità, diventando, quindi, un concreto ausilio anche alle famiglie. Lo sport è amore, è passione, perché mobilita, attraverso i praticanti a tutti i livelli e gli appassionati, sentimenti positivi di milioni di persone. Lo sport è volontariato, perché coinvolge un gran numero di persone che, gratuitamente, prestano la loro attività affinché diversi settori sportivi possano operare e svilupparsi. E senza di loro alcune discipline non sarebbero cresciute ai livelli attuali. Lo sport è anche economia, collegata sia alla pratica sportiva che all'attività dilettantistica che all'attività dello sport spettacolo. E questo avviene non solo nel calcio. Oggi l'importanza dell'indotto dell'economia dello sport, degli *sponsor*, delle trasmissioni sportive appare evidente anche per molti degli sport che una volta venivano considerati minori. Lo sport è stare insieme. Abbiamo visto quale importanza ha il ruolo dell'associazionismo, che ha dovuto affrontare il triste periodo delle chiusure pandemiche e delle limitazioni di molte attività, incluse quelle sportive. Il riconoscimento della dignità dell'attività sportiva in Costituzione potrà dare un ulteriore impulso all'iniziativa legislativa ordinaria e faciliterà l'operosità delle tante associazioni sportive. Lo sport è formazione e cultura per i nostri giovani, perché insegna l'inclusione, insegna il valore dell'amicizia, insegna il sentimento di gruppo, insegna il rispetto dell'avversario, insegna il sacrificio e la dedizione per ottenere i risultati, insegna il valore del merito, insegna la solidarietà, insegna il rispetto per la disabilità, insegna a ripartire dopo una sconfitta. Come vedete, molti dei valori che esprime lo sport sono già presenti in Costituzione. È ora che ci entri lo sport stesso ed è per questa ragione che annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. Presidente, signori del Governo, onorevoli senatrici e senatori, all'indomani delle elezioni il MoVimento 5 Stelle ha detto che sarebbe stato una forza di opposizione ferma e intransigente, ritenendo sbagliate le ricette

che avremmo ritenuto potessero andare incontro al Paese, alle famiglie, soprattutto ai nostri giovani. Pertanto, coerentemente con quello che dicemmo, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla modifica dell'articolo 33 della Costituzione in materia in Ricordo a tutti, *in primis* a me stesso, che veniamo da due anni di pandemia, due anni difficili, dove per i nostri ragazzi, per i giovani, la normalità era il *lockdown*, erano la paura del contagio e il distanziamento sociale; un'emergenza che ha lasciato profonde cicatrici, soprattutto nelle giovani generazioni, e ha portato a un forte isolamento, a solitudine e stress nei ragazzi, con un cambio completo della loro vita quotidiana. Lo sport, in quei momenti, è stato centrale e rappresenta una chiave fondamentale, proprio in questo momento, per ripartire. Secondo studi recenti molto molto importanti chi vive lo sport lo vive come una valvola di sfogo. Le giovani generazioni riescono a ricaricarsi dallo stress e dalle ansie che accusano dalle fatiche scolastiche e dalla vita quotidiana. Quindi ogni misura che sarà al fianco dei giovani

di avere accesso facile allo sport. Il 50 per cento di questi giovani crede, inoltre, che nelle strutture scolastiche non ci siano campi sportivi idonei,

Lo studio va nello specifico: molti sono i problemi, tra cui ragioni di studio, allenamenti troppo duri, problematiche con gli allenatori, tempo libero praticamente inesistente oppure competizione eccessiva. Ci sono però alcuni punti, che toccherò più avanti, che riguardano le distanze degli impianti sportivi e il costo per praticare lo sport: accedere alle strutture sportive per fare sport ha un costo importante. Oggi - secondo me di diritto - all'interno della Costituzione, all'articolo 33, nel quale si parla di arte, di scienza, di insegnamento, di scuola, di diritto, di istruzione, di cultura e di università, si inserisce una frase, che cito: «La Repubblica riconosce» - e lo sottolineo - «il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». valore educativo; sì, perché lo sport è questo. Lo sport insegna ed educa le persone; le educa quando si impegnano in prima persona per raggiungere un obiettivo; ma le educa anche quando si lavora in gruppo, quando si capisce che una dinamica si fa con più persone per raggiungere degli obbiettivi. Lo sport educa anche a curare la propria forma fisica, il proprio aspetto, il proprio corpo in maniera attenta

chi è in difficoltà e gli stiamo precludendo di fare sport in questo momento. Senza calcolare poi i tagli alla scuola che saranno pesantissimi da qui in avanti. avanti. Abbiamo poi dei modelli che ci vengono raccontati, che vengono narrati; il *mainstream* parla spessissimo di personaggi sportivi. Se voi chiudete gli occhi e pensate ai campi da gioco dei Paesi

Ringrazio anche chi era al Governo con noi quando ha dato la possibilità a Giuseppe Conte di eliminare il gioco d'azzardo *(Applausi)* dalla promozione e dai programmi televisivi, dai luoghi pubblici e da tutti gli spazi

che sui campi da giochi e dentro le palestre, a titolo gratuito, si prendono cura del benessere dei nostri figli e li accompagnano in un percorso di crescita. Ecco, anche a nome di queste persone che tutti i giorni aiutano i nostri figli a crescere, dichiaro, a nome del MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Questo comma, inserito nell'articolo 33 della Costituzione, è di una straordinaria bellezza e racchiude in sé una quantità infinita di valori e significati. per me, quindi, un grande onore accingermi, a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, a dichiarare il voto favorevole sul disegno di legge costituzionale al nostro esame. Quali sono i valori e significati che riconosciamo oggi in Costituzione? Cosa è lo sport? È salute, integrazione, socializzazione e riscatto, amicizia, passione, espressione delle migliori energie e talenti, capacità di concentrazione, sofferenza e sforzo per raggiungere un obiettivo. È imparare a cadere e rialzarsi, a riconoscere i meriti altrui e i propri limiti. È coraggio, etica - nessuno ti regala nulla - lealtà, correttezza, rispetto delle regole dell'avversario. È imparare a conoscere se stessi e i propri limiti. È gioia, ma anche sofferenza, sacrificio costante e sforzo per migliorare con fatica ogni giorno. superare la paura del gesto atletico e della competizione con gli altri. È equilibrio tra mente e corpo. È libertà dell'essere. È pura bellezza. È tutto questo e tanto altro ancora. Tutti questi sono insegnamenti di valore incommensurabile per la vita di ogni uomo e per la crescita dei nostri ragazzi. C'è un mondo meraviglioso che ruota intorno allo sport. Conosciamo tutti le grandi società calcistiche e le poche altre realtà attorno a cui ruotano interessi economici rilevantissimi. Ma il mondo dello sport è fatto soprattutto da un'infinità di società sportive, di istruttori, di allenatori, di tesserati, di genitori e tanti volontari che, con dedizione e straordinaria passione, svolgono per i nostri ragazzi un lavoro che non ha prezzo. Lo Stato deve investire molto di più su questa realtà dal punto di vista sia del finanziamento alle associazioni sportive che di quello delle infrastrutture. Tutto ciò che ha a che fare con l'attività sportiva ha, inoltre, dei risvolti importantissimi non solo per gli aspetti che ho prima elencato, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. È di dominio comune, in primo luogo, il fatto - comprovato scientificamente con dati statistici ad ogni livello - che l'attività sportiva incide sul miglioramento delle condizioni fisiche, sulla prevenzione della malattia e funge da elemento deterrente contro l'abuso di sostanze e il mondo della criminalità, ingenerando importantissimi risparmi sui costi della sanità e per il sistema giustizia. Lo sport, però, non si limita a ingenerare risparmi, ma significa anche aumento del PIL. Vengo da una Regione meravigliosa, la Valle d'Aosta, che madre natura ha creato come palestra a cielo aperto. Noi quindi sappiamo bene che sport significa anche turismo e, quindi, economia. Tutto questo ha aiutato a sviluppare una sensibilità molto forte da parte non solo dei cittadini, ma anche dell'amministrazione a tutti i livelli nei confronti dello sport, e le politiche attive in tale direzione sono assolutamente virtuose. I dati statistici, però, fotografano una realtà italiana non omogenea, con grandi disparità tra le diverse zone e realtà e, quindi, lo Stato deve fare molto di più di ciò che è stato fatto finora. Sono convinta che oggi sia stato fatto un primo, importantissimo passo per la valorizzazione dello sport, a cui faranno seguito tanti altri interventi concreti a molteplici livelli. Come ho già detto in Commissione, spero che una particolare attenzione venga data dal Ministro per lo sport, in raccordo con il Ministro per l'istruzione, al mondo della scuola, dove ancora non si fa abbastanza per spingere i nostri ragazzi ad approcciarsi allo sport vero e proprio e non solo a una semplice attività fisica. Il vero cambiamento non può non passare anche attraverso un approccio - molto più elastico di quanto ad oggi non si abbia da parte del mondo scolastico - con chi svolge attività sportiva a livello agonistico. Nessun ragazzo, se meritevole e studioso, dovrebbe mai essere posto davanti alla scelta tra la propria istruzione e l'attività agonistica, che spesso comporta delle assenze giustificate dalle competizioni. Molto spesso i migliori studenti sono proprio quelli che si dedicano con grandi sacrifici agli allenamenti, strutturando la propria giornata su studio e sport, con tempo libero quasi nullo e con una capacità di concentrazione elevata, sviluppata dalla necessità di fare i compiti a casa e preparare interrogazioni e compiti in classe senza concedersi tempi morti davanti alla TV, attaccati ai *social* o altro. Bisognerebbe rendere strutturali tali possibilità, come avviene in molti altri Paesi, e con una elasticità che non può essere delegata alla sola sensibilità personale da parte dei tanti professori eccezionali che si rendono conto dell'importanza, per i ragazzi, di poter portare avanti scuola e sport contemporaneamente. Fiduciosa della volontà di questo Governo e in particolare del Ministro di lavorare in tale direzione, come già annunciato, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

molto volentieri, a nome del Gruppo Partito Democratico. L'ho fatto diverse altre volte, perché l'*iter* di questa riforma è stato complesso e lungo - poi spiegherò perché e lo faccio per esprimere un convincimento e anche un auspicio. Il convincimento che esprimo ha a che vedere con l'importanza della riforma, che eleva a valore costituzionale il Ministro - è importante sul piano della salute mentale e fisica delle persone; è importante in termini di coesione sociale; è importante sul piano anche morale, della crescita caratteriale delle persone, della socializzazione e dell'apprendimento su come costruire relazioni umane improntate alla correttezza e durature. Noi facciamo quindi il nostro dovere approvando questa riforma. Ci auguriamo che quello odierno sia l'ultimo passo del Senato verso l'approvazione definitiva (come sappiamo è la seconda lettura). terzi dei componenti l'Assemblea e che lo stesso avvenga alla Camera, in modo da non dover attendere tre mesi per la promulgazione della riforma e per poter salutare una sua immediata entrata in vigore. Contemporaneamente sappiamo che questa riforma è un punto di partenza e non un punto di arrivo: anche questo concetto è stato ricordato nel dibattito che abbiamo svolto. È un punto di partenza nel senso che dà una spinta al legislatore, rende solenne l'importanza dello Sport all'interno della nostra società. Poi però, perché davvero l'accesso all'attività sportiva diventi più largo, perché davvero il diritto allo sport diventi un diritto per tutti effettivamente esercitabile, occorre - lo dico in particolare al Governo che vengano approntate risorse sufficienti, che tutto il vasto mondo dello sport a tutti i suoi livelli possa contare su infrastrutture adeguate e svolgere il proprio lavoro con serenità e senza scarsità di mezzi. Noi vogliamo che questa riforma faccia la differenza per tutto lo sport a tutti i livelli: per lo sport amatoriale come per quello svolto a livello agonistico, per quello professionistico come per quello dilettantistico, per lo sport di base come per lo sport di vertice. Noi che portiamo avanti questa riforma nella società c'è un'aspettativa che non possiamo deludere. Se ci limitassimo a cambiare l'articolo 33 della Costituzione senza far seguire a questo atto delle scelte concrete, compiremmo un errore. Concludo il mio intervento - desidero essere molto breve ricordando che l'*iter* di questo provvedimento è tipicamente unitario. È cominciato nella scorsa legislatura. Abbiamo scritto la norma nella sua formulazione attuale all'interno della Commissione affari costituzionali che presiedevo

di riprendere quella formulazione senza modifiche, per arrivare speditamente al risultato e credo che ci possiamo riuscire. Alla luce di questo fatto, proprio perché oggi arriviamo dove saremmo arrivati anche nella scorsa legislatura se non ci fosse stata l'interruzione anzitempo e non ci fossero state le elezioni anticipate, mi sento di invitare a una maggiore cautela gli esponenti della maggioranza che, come la senatrice Biancofiore, hanno teso a fare di questa riforma l'oggetto di una vanteria e di una rivendicazione di parte. *(Applausi).* È sbagliato, oltre che fattualmente non corrispondente alla verità.

quanto è stato detto corrisponde a realtà - questo è un lavoro di sintesi politica partito nella scorsa legislatura, quando si erano consumati i tre passaggi ed è mancata soltanto l'approvazione finale. Credo che il momento sia assolutamente solenne e non soltanto perché perché è doveroso quando si va a toccare la nostra Carta costituzionale. Il momento è solenne perché esiste un mondo fatto di milioni di praticanti che lo aspetta da tanti anni. questa occasione di rendere giustizia, merito e dignità a tutti coloro che hanno portato avanti il nostro mondo sportivo possa finalmente conoscere, con l'impegno di tutti, la sua consacrazione con il riconoscimento all'articolo 33 della Costituzione. Credo che non ci sia nessuno che voglia rivendicare protagonismi di parte, ma con orgoglio tutti possano dire quello a cui per anni si è lavorato e aspirato. Anch'io voglio dire che a destra c'è stata sempre una grande sensibilità nei confronti di questo mondo. Voglio ricordare che la prima proposta di legge costituzionale per il riconoscimento del valore dello sport fu presentata a metà degli anni Novanta dal compianto senatore Giulio Maceratini all'epoca Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale proprio in questo ramo del Parlamento. È doveroso, da parte mia, ringraziare, oltre che tutti i parlamentari che hanno espresso un voto favorevole nei due rami del Parlamento,

per trovare l'intesa che è conclamata in questo progetto di legge. Desidero, quindi, veramente ringraziare in maniera accorata il senatore Parrini, che era Presidente della Commissione affari costituzionali nella scorsa legislatura. Voglio ringraziare il nostro presidente Alberto Balboni, che è anche relatore in Aula. Voglio ringraziare l'onorevole Urzì, che è stato relatore alla Camera dei deputati. E voglio anche ringraziare coloro che nella scorsa legislatura, nel Comitato ristretto nella Commissione affari costituzionali, hanno svolto il lavoro di confronto - in particolare il senatore Claudio Barbaro e il mio Capogruppo Lucio Malan che oggi ci consentono, in virtù di quel lavoro già avviato, di essere qui per questo voto finale che - ribadisco dà dignità, riconoscimento e piena cittadinanza nella nostra società al mondo straordinario dello sport, che rappresenta uno dei racconti migliori della nostra Patria. Si è voluto riconoscere l'attività sportiva in ogni sua forma, e quindi non soltanto lo sport competitivo, quello dei risultati, quello dei grandi campioni, che pure ci riempie di orgoglio e gioia e ci fanno sentire più italiani nei momenti delle vittorie, ma anche quello di tutti coloro che praticano lo sport perché intimamente convinti che rappresenti uno strumento eccezionale, lo strumento migliore per realizzare tanti obiettivi sociali; per fare in modo che in maniera trasversale, dai giovani ai più anziani, attraverso lo sport si possa costruire un modello nuovo e più positivo di comunità nazionale. Per quanto riguarda i giovani, infatti, il Ministro sa benissimo che lo sport rappresenta l'arma migliore per tenerli lontani dalle devianze e da alcuni stili di vita di strada che rappresentano un grave rischio e un grave momento di socialità che viene poi agli onori della cronaca. Rappresenta lo strumento attraverso il quale realizziamo anche obiettivi di sanità pubblica, perché - diciamolo - lo sport fa bene e aiuta a tenere coinvolti, vivi e attivi anche coloro che hanno qualche anno in più, ma non rinunciano ad uno stile di vita sano. Noi siamo convinti che le scelte che sono state fatte dal nuovo Governo e dal presidente Meloni, che peraltro ha voluto inserire nel programma elettorale elettorale il riconoscimento dello sport in Costituzione, insieme a tante altre iniziative che il Ministro ha già avviato, sono state scelte giuste. Innanzitutto,

si è voluto fare in modo che questo aspetto di grande importanza sociale fosse al centro e non più marginale nelle politiche di sviluppo sociale di un Governo. La scelta del Ministro parla di un uomo di sport, un uomo competente che ha dimostrato nei suoi precedenti incarichi di sapere di che cosa parla e che cosa fa. fa. Sono d'accordo con tutti gli interventi che ho ascoltato: deve essere un punto di partenza, però, lo ricordo a tutti noi,

e a tutti, naturalmente annunciando il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, le parole che furono pronunciate da un indimenticato presidente del CONI, Giulio Onesti, quando molti anni fa disse: «Una società moderna deve dare ai giovani la possibilità di conoscere lo sport facendoli uscire dalle gabbie di cemento e di ferro in cui li hanno rinchiusi gli errori dei grandi. E ci sembra opportuno che il privilegio di pochi divenga anche in Italia il diritto di tutti». Con questo voto tutti insieme possiamo consegnare queste parole alla storia e e aprire una nuova era per questo mondo straordinario che ha dato tutto alla nostra Nazione.

apre una nuova finestra"). Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»

ma vi chiedo la gentilezza di lasciarci proseguire con l'andamento dei lavori. Ha

Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Promossa dal comitato internazionale per la Giornata contro l'omofobia e la transfobia, questa giornata è riconosciuta e celebrata dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite. L'obiettivo della giornata odierna è promuovere e coordinare eventi internazionali di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia, della bifobia, della transfobia, e possibilmente anche della maleducazione...

che quest'Assemblea, scegliendo di discutere oggi di questa mozione in maniera unitaria, sta realizzando un grande evento di sensibilizzazione. La scelta della data del 17 maggio non è certo casuale. È infatti in questo giorno che, nel 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità rimosse l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali, specificando che non esiste alcuna devianza e alcuna patologia, ma che l'orientamento sessuale fa semplicemente parte dell'identità di ogni essere umano. Ebbene, nonostante siano passati trentatré anni da quella declassificazione, il cammino per l'affermazione della parità dei diritti delle persone *gay*, lesbiche, transgender, bisessuali o non binarie è ancora impervio e lungo. Ancora oggi sono ben 71 i Paesi nel mondo che hanno leggi punitive contro l'omosessualità e gli orientamenti sessuali. Proprio il 21 marzo scorso il Parlamento dell'Uganda ha approvato una delle leggi più severe, che configura come reato l'attività sessuale consensuale tra adulti dello stesso sesso, prevedendo addirittura la pena di morte in alcuni casi e introducendo il carcere fino a vent'anni per le persone che si dichiarano omosessuali. Purtroppo, però, è praticamente tutto il continente africano a non essere un luogo sicuro; non è esattamente il miglior luogo dove nascere se si è *gay*, lesbiche o transgender. In Mauritania, Sudan, Nigeria settentrionale e Somalia meridionale è prevista la pena di morte - come riportano i dati di Amnesty International - anche in altri Paesi l'omosessualità è considerata un reato ed è punita con il carcere. Le leggi più severe sono in Gambia, Sierra Leone e nell'area centro africana (Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia), dove è previsto persino l'ergastolo. Ci sono poi Stati, come l'Eritrea e il Sud Sudan, in cui le persone a causa del loro orientamento sessuale possono subire condanne dai sette ai La Libia e il Camerun prevedono la detenzione fino a cinque anni, il Marocco la detenzione fino a tre anni, così come in Ghana, Guinea, Togo e Tunisia. In Algeria e Ciad il reato è punito con due anni di carcere, in Liberia e Zimbabwe con uno; in molti dei Paesi menzionati sono previste anche sanzioni economiche e multe in aggiunta alla detenzione. La situazione non è certo migliore in molti Paesi arabi: in Iran è prevista la flagellazione, in Arabia Saudita la lapidazione, negli Emirati Arabi Uniti la pena di morte. di morte. La situazione è drammatica anche in Afghanistan, soprattutto dopo il ritorno al potere dei talebani. Il motivo per cui oggi siamo qui è che, il 18 dicembre 2008, 66 Stati hanno sostenuto una dichiarazione dinanzi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, esortando gli Stati ad adottare tutte le misure necessarie, in particolare legislative o amministrative, per garantire che l'orientamento sessuale e l'identità di genere non possano in alcun caso costituire la base per sanzioni penali, in particolare esecuzioni, arresti o detenzioni. Il 4 maggio 2015 l'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha raccomandato agli Stati di rivedere il loro diritto penale al fine di sopprimere i reati relativi a comportamenti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso, ordinare una moratoria immediata sulle pertinenti azioni penali e cancellare tali reati dai casellari giudiziari delle persone condannate. Ecco dunque perché siamo qui ed ecco perché voglio, innanzitutto, ringraziare tutti voi, colleghe e colleghi di tutti gli schieramenti e Gruppi politici presenti qui dentro. So bene che, per raggiungere questo testo unitario, tutti abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa che riteniamo importante rinunciare all'orgoglio politico di differenziarci. Abbiamo rinunciato a qualcosa di importante, ma l'abbiamo fatto per raggiungere qualcosa di fondamentale: l'impegno del Governo a sostenere, nelle competenti sedi istituzionali europee ed internazionali, un'ampia coalizione di Stati per promuovere la depenalizzazione universale dell'omosessualità, a garanzia del rispetto dei diritti umani universali in cui tutte e tutti noi crediamo. Voglio ringraziare infine tutte le associazioni che si battono per i diritti LGBT in Italia, perché senza il loro sostegno questo Senato non avrebbe raggiunto oggi questo risultato.

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, ribadiamolo quindi: il 17 maggio di ogni anno si celebra in tutta Europa la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, per denunciare ogni forma di violenza legata all'orientamento sessuale. una data con un forte valore simbolico e storico: è il giorno in cui, nel 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità rimosse l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali, specificando che non esiste nessuna devianza e patologia, ma che l'orientamento sessuale fa semplicemente parte dell'identità di ogni essere umano. La prima considerazione che viene in mente è che la maggior parte di noi è nata ed è cresciuta in un mondo che considerava l'omosessualità una malattia mentale. Questo ci dà la misura del cammino che, come società, dobbiamo fare per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione. Sul piano internazionale (quello a cui si riferisce questa mozione), trent'anni dopo quella declassificazione il cammino per l'affermazione della parità dei diritti delle persone omosessuali è ancora più lungo e difficile. Ad oggi 71 Paesi hanno leggi punitive contro l'omosessualità. Da ultimo, il parlamento dell'Uganda ha approvato uno dei più severi disegni di legge al mondo, una legge fermamente condannata dal Parlamento europeo, una legge che Amnesty International ha definito spaventosa, ambigua e formulata in modo vago. Questo provvedimento stabilisce pene atroci per i reati legati all'omosessualità, sino ad arrivare alla pena di morte per omosessualità aggravata. Prevede anche l'obbligo di denuncia delle relazioni omosessuali da parte della famiglia e della comunità. In Nigeria le persone omosessuali vengono condannate alla lapidazione. Sicuramente, come abbiamo ribadito, il continente africano è quello con leggi più severe, con pene che variano dalle condanne dai sette ai dieci anni fino alla condanna all'ergastolo e fino alla pena di morte. La situazione non è migliore in Afghanistan, dove è prevista la flagellazione e la lapidazione. Anche laddove il codice penale non prevede formalmente la pena di morte, non è raro vedere uomini e donne uccisi dalle milizie o essere condannati dai giudici in base alla *sharia*, come in Iraq. Capita anche che le persone siano condannate per il semplice fatto di aver supportato i diritti della comunità LGBTQIA+. In Iran, due donne sono state condannate a morte in quanto colpevoli del reato di corruzione sulla terra, ai sensi dell'articolo 286 del codice penale islamico. Senza considerare tutte quelle persone impiccate persone impiccate in piazza, la cui colpa era quella di amare qualcuno del proprio sesso. In un contesto internazionale dove si fa fatica ad affermare i diritti delle persone omosessuali, cosa possiamo fare? Come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di chiederci quale sia il nostro ruolo in tutto questo e in che modo il nostro Paese può agire nel contesto internazionale. Non possiamo di certo stare a guardare e non possiamo far finta che questi avvenimenti siano lontani e siano a noi estranei, perché, in questi casi, in questi casi, stare a guardare senza condannare queste brutalità equivale ad avallarle. Abbiamo l'obbligo etico di condannare. Cosa possiamo fare? Oggi sicuramente una cosa possiamo farla. Oggi è un'ottima giornata. Oggi è la giornata in cui quest'Aula si impegna a proteggere le persone omosessuali da qualunque forma di violenza anche prevedendo, in accordo con altri *partner* internazionali, delle attività diplomatiche volte a modificare la legislazione di quei Paesi che annoverano nei propri ordinamenti dei trattamenti non rispettosi della dignità umana, perché è di questo che stiamo parlando: agire sul piano internazionale con passi concreti, piccoli, certo, ma costanti.

pensando a Paesi in cui la libertà sessuale è negata, dobbiamo avere l'umiltà di rivolgere lo sguardo anche alle nostre comunità, anche alla nostra società, dove l'orientamento sessuale non è reato, è riconosciuto quale espressione dell'identità personale, ma dove, tuttavia, non sono estranei gli episodi di discriminazione, talvolta di violenza morale e fisica. allora, questa occasione per riflettere anche sulle forme di diffusione di una cultura di libertà e di non discriminazione, su cui anche il nostro Occidente non può considerarsi arrivato. La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, che tutti noi conosciamo come "Commissione Segre", di cui ho l'onore di fare parte, può costituire una importante sede di confronto per valutare l'individuazione di una strategia comune a tutte le forze politiche. La mozione di oggi, sottoscritta in maniera trasversale, è un ottimo segnale, perché questo compito di intervenire a livello internazionale non può e non deve essere il manifesto di questo o di quel partito. La tutela dei diritti umani è patrimonio di tutte le forze politiche e democratiche e deve essere un minimo comune denominatore di tutti coloro che si riconoscono nei valori della nostra Costituzione. Con la mozione in oggetto chiediamo che il Governo si impegni a sostenere, nelle competenti sedi istituzionali internazionali, una ampia coalizione di Stati per promuovere la depenalizzazione universale degli orientamenti sessuali, a garanzia del rispetto dei diritti umani universali. Lo chiediamo con forza e con convinzione, consapevoli di dover vigilare sul contrasto ad ogni forma di discriminazione. *(Applausi)*.

mondiale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Ovvero potremmo dire che è la giornata mondiale in cui ci accorgiamo che l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono dei diritti umani e che come tali vanno riconosciuti.

mondo questo principio non sia ancora entrato, non solo nel comportamento magari dei Governi, ma anche nell'orientamento comune. Molte sono, inoltre, ancora le forme di tortura, perché in tal modo andrebbero definite - e sono riportate nella mozione - le reazioni che ci sono, le forme di

Circola l'odio nei confronti di coloro che sono diversi e viviamo come differenti; circola nei *social*, nel linguaggio pubblico e devo dire che spesso sottovalutiamo come nel discorso pubblico, anche di persone importanti che rappresentano opinioni o istituzioni nel nostro Paese, quando poi si parla per pregiudizi si determinano dei danni dal punto di vista del rispetto e del riconoscimento del mondo. Quindi in realtà si cade esattamente nelle forme di persecuzione, di omofobia, di bifobia e transfobia. allora dobbiamo interrogarci sul perché succede tutto questo e sul perché abbiamo ancora difficoltà a rispettare chi è diverso da noi stessi, perché, nel rifletterci nell'altro, abbiamo bisogno di avere la conferma che è uguale e non gli riconosciamo eguaglianza. È una paura che ci fa determinare poi dei comportamenti che sfociano ancora nell'esistenza di forme di violenza e di oppressione nei confronti di chi è diverso da noi. Peraltro, come abbiamo visto, giustamente chiediamo agli altri Paesi di rispettare i diritti, ma tuttora non abbiamo una legge che condanni l'omofobia, la bifobia e la transfobia: non siamo riusciti a farla. In questi giorni abbiamo scoperto che, tra le tante paure che abbiamo rispetto a quelli differenti da noi, abbiamo anche la paura di guardare in faccia i bambini e le bambine e chiediamo loro che origine hanno e non gli riconosciamo uguaglianza di diritti, nonostante siano appunto dei bambini e delle bambine. allora ad avere un problema di diversità perché, se non riusciamo ad ammettere che un diritto è tale se è universale e che un diritto non è un dovere, nel momento in cui si riconoscono a tutti i diritti, non ci si obbliga a comportamenti che magari non sono nelle nostre corde, noi continuiamo a confondere questi due aspetti. Pensiamo che riconoscere un diritto a chi è diverso diventi in qualche modo un vincolo per i nostri comportamenti; ma allora abbiamo un problema, sia con la definizione dei diritti umani, ma direi - come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica in queste ore - anche con l'articolo 3 della Costituzione *(Applausi)*, che ci dice che dobbiamo rimuovere tutti gli ostacoli affinché le persone siano in uguaglianza. in uguaglianza. Poco fa abbiamo votato, e l'Aula ha grandemente festeggiato, l'inserimento dello sport nella nostra Carta costituzionale. Ebbene, dobbiamo sapere che, anche se parliamo di sport, ci sono persone che, nel percorso di transizione o al completamento del loro percorso di transizione, si vedono negare il diritto e la libertà di continuare a fare attività sportiva, perché c'è chi ha paura di riconoscere che ci sono delle differenze nei percorsi che vengono fatti, che non vincolano noi, ma che vanno riconosciuti. modo qualche volta abbiamo paura di riconoscere che, se c'è un percorso di transizione, questo non solo ha degli effetti sui cosiddetti diritti civili, ma ha dei concreti effetti sui diritti sociali. Dobbiamo dirci che, se si è persone trans, è più difficile avere un lavoro? Possiamo dirci che, se si è persone trans, è più difficile avere il riconoscimento del proprio sentire e, quindi, l'uso dell'*alias*, ma si è costretti a lunghi percorsi? In tutti questi casi qual è la ragione che lo determina, se non la nostra paura di riconoscere comportamenti diversi come altrettanto legittimi? E allora credo che in questo giorno dobbiamo guardare al resto del mondo, ma guardare anche a come siamo noi stessi, a come la separazione che troppo spesso si fa tra diritti civili e diritti sociali in realtà non veda come il fatto che non si riconoscano a tutti gli stessi diritti ha effetti sul terreno civile, ma anche sul terreno sociale, del lavoro e della propria convivenza.

sessuali, dell'identità di genere e della libertà delle persone, ma anche di come tutto questo poi si traduca nel fatto che si vogliono marginalizzare ed emarginare persone che avrebbero invece diritti. Permettetemi di sottolineare che in quel lungo elenco ce ne sono alcuni di Paesi che parlano anche a noi, che parlano anche alle scelte che sono state fatte negli anni dalle grandi coalizioni di cui noi facciamo parte e che, forse, hanno avuto l'esito più infausto che si poteva avere. Io non posso in questa giornata non rivolgere un pensiero agli afgani, alle donne afgane e alle persone LGBTQIA+ in Afghanistan perché sono le vere vittime di quell'abbandono che abbiamo determinato nell'agosto di qualche tempo fa. Così come non possono rivolgere un pensiero ai ragazzi e alle ragazze dell'Iran che continuano, nonostante su molti di loro sia caduto il silenzio, il silenzio, una lotta per la loro libertà, che è fatta innanzitutto esattamente della stessa cosa: riconoscere il loro libero diritto di essere come vogliono essere e non avere condizionamenti e vincoli. Eppure, in quel Paese, di giorno in giorno aumentano le condanne a morte e sono tutte condanne a morte di persone che hanno semplicemente cercato di affermare un loro diritto. Faccio questo ragionamento perché noi giustamente chiediamo al Governo di sostenere nelle sedi istituzionali europee ed internazionali gli orientamenti che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i responsabili dei diritti umani hanno sostenuto e, quindi, il fatto che ci sia la promozione della depenalizzazione universale delle condotte relative ai rapporti consensuali tra persone adulte dello stesso sesso e la garanzia del rispetto dei diritti umani universali. Vorrei dire però al Governo che serve una cosa in più, che è quella di avere il coraggio di dire che la qualità del riconoscimento delle libertà delle persone è parte della politica internazionale: che qualche volta bisognerebbe avere il coraggio di non considerare sicuri Paesi che magari sono alleati, ma poi concretamente nel loro territorio esercitano la repressione. Cosa è un Paese sicuro? Forse dobbiamo definirlo esattamente alla luce del fatto che non c'è Paese sicuro se le persone non sono libere di esprimere il loro orientamento sessuale, la loro identità di genere e di venir riconosciute come persone, di cui non si deve aver paura e tantomeno che si possono perseguitare.

Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che questa sia una di quelle giornate nelle quali dobbiamo essere particolarmente contenti e direi fieri ed orgogliosi di far parte del mondo libero, di vivere in un Paese solidamente democratico, che ha a cuore la libertà dei singoli cittadini in tutti gli ambiti in cui questa libertà si può esprimere e concretizzare. La mozione che i Gruppi parlamentari hanno proposto all'approvazione di quest'Aula - ed è davvero un ottimo segnale che sia un atto unitario - ci ricorda che cosa accade fuori dai confini dell'Europa e spesso a poca distanza dai nostri confini. Dovremmo ricordarcene sempre. Dovremmo ricordarcene quando le battaglie di libertà che si combattono in tante parti del Pianeta escono fuori dai radar della nostra agenda; dovremmo ricordarcene quando, troppo spesso, noi stessi siamo inclini a sottovalutare o addirittura in alcuni casi a disprezzare la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra identità e magari non sottoponiamo altre culture allo stesso vaglio critico; dovremmo ricordarcene quando mettiamo in dubbio la nostra collocazione nel mondo. Questa Giornata ci ricorda che il corpo è fondamentale e che la libertà riguarda ognuno di noi come persona e quindi, in primo luogo, riguarda il nostro corpo. Abbiamo ricordato in altre occasioni come sia importante la libertà delle donne in Iran e in Afghanistan - è stato ricordato in quest'Aula anche in questo momento - tanto che, per difendere la semplice scelta di non indossare il velo o di sciogliere i capelli, le ragazze e le donne sono disposte a lottare fino a rischiare la vita. Ricordiamo oggi che è fondamentale ovunque la libertà sessuale delle persone, di ogni persona adulta e consenziente, qualsiasi sia la sua inclinazione, qualsiasi sia il suo orientamento, qualsiasi sia la persona che decide di amare, e che dobbiamo lottare contro ogni discriminazione, violenza e pregiudizio in questo campo. Questa libertà non dobbiamo soltanto tenercela stretta, ma ogni giorno difenderla nel nostro Paese e nel mondo: questo Governo si impegna in tal senso con decisione. Abbiamo fatto un lungo percorso sulla strada della libertà delle scelte affettive e sessuali, se confrontiamo la situazione che viviamo oggi con quella di pochi decenni fa: è un fatto consolante su cui bisogna continuare a lavorare, perché è importante avere anche la piena consapevolezza del cambiamento culturale che è avvenuto, per poterlo valorizzare, ampliare e difendere; perché lungo la strada della libertà si può e si deve sempre fare di più; perché in Italia ogni persona, oltre ad essere libera, deve anche sentirsi pienamente libera. Il Il Governo esprime parere favorevole sulla mozione sul contrasto all'omofobia n. 47, a firma dei senatori Maiorino, Malan, Bazoli, Romeo, Scalfarotto, Ronzulli, Unterberger, Biancofiore e De Cristofaro.

17 maggio, ricorre la Giornata internazionale contro l'omofobia. Da quest'Aula si leva un messaggio di giustizia e di equità sociale, credo senza precedenti. Il 17 maggio è una giornata che ha un forte valore simbolico e storico. Infatti, trentatré anni fa l'Organizzazione mondiale della sanità rimuoveva l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Essere omosessuali non è una malattia; essere omosessuali non è - e non può essere, neppure - considerato un crimine. In questo mio intervento vorrei richiamarmi alle parole di sua santità Papa Francesco, che più volte nel corso del suo pontificato ha richiamato la cultura del rispetto dell'altro. Ogni persona ha dignità. Storica la sua prima frase pronunciata nel 2013 all'alba del suo pontificato: «Chi sono io per giudicare?» A gennaio scorso abbiamo ascoltato tutti con profonda attenzione il suo appello per la depenalizzazione dell'omosessualità in tutto il mondo. nonostante siano passati trentatré anni da quel 17 maggio, ancora oggi settantun Paesi del mondo hanno leggi punitive contro gli orientamenti sessuali. In Uganda - ma è solo un esempio - due mesi fa il Parlamento ha approvato una legge che punisce con vent'anni di carcere le persone che si dichiarano omosessuali, e introduce ulteriormente la pena di morte in caso di determinate aggravanti. non succede solo in Uganda, purtroppo: in Africa situazione simili si registrano anche in Mauritania, in Sudan, in Nigeria, in Somalia. In Afghanistan, ad esempio, dopo il ritorno al potere dei talebani, vige la legge la legge A causa della *sharia*, i diritti delle persone vengono quotidianamente calpestati. Morire schiacciati da un muro alto tre metri o, in alternativa, essere lapidati: è questa la pena di morte prevista. Apro una breve parentesi: a Kabul e in tutto il Paese, secondo le denunce di autorevoli fonti (tra cui Amnesty International), il Governo talebano ha messo in campo tutta una serie di misure contro le donne e persino le bambine: per loro è vietato andare a scuola, in palestra, negli *hammam* o in altre parti. Per loro, donne e bambine, è vietato - in una parola - vivere; anche per le persone omosessuali purtroppo è ancora così. I diritti inalienabili appartengono a tutti. Ce lo dice a chiare lettere la nostra bellissima Costituzione. Faccio riferimento all'articolo 3 della nostra Carta, che prevede il principio dell'uguaglianza. Al primo comma si stabilisce il concetto di uguaglianza formale, ma il secondo comma, che introduce il concetto di eguaglianza sostanziale (su cui mi soffermerò a breve), è il cuore del principio che sta alla base di tutto: la pari dignità tra le persone. Ciascuno di noi ha attitudini diverse, talenti diversi; sappiamo innanzitutto di essere differenti. Allora la domanda è: siamo davvero uguali? davvero uguali? Assolutamente no. Ognuno di noi ha il proprio profilo originale, ha un bagaglio che va a influire nel percorso della propria vita. L'uguaglianza tra le persone è basata sul valore della dignità: la pari dignità di cui parla la nostra Costituzione. Ogni persona è unica e irripetibile. Occorre sviluppare gli anticorpi contro una cultura che considera alcune vite di serie A e altre di serie B. Siamo pronti: su certi temi dobbiamo essere tutti uniti, non è il tempo della retorica sterile; siamo per la cultura del rispetto dell'altro più volte richiamata dal Pontefice. Questa cultura del rispetto dell'altro va tradotta però in azioni concrete. La parola chiave è proprio questa: rispetto. Non basta, infatti, la sola tolleranza; serve il rispetto, che significa riconoscere l'altro non come estraneo, ma come parte di sé stesso. rispetto, perché nessuna appartenenza rinunci alla propria identità. Per questo ho citato entrambi i commi dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Il secondo comma di questo articolo, infatti, afferma chiaramente che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva uguaglianza. I diritti sono di tutti, nessuno escluso.

Questa è la nostra cultura politica e ne siamo fieri. Chiaramente siamo perché ci siano una mamma e un papà, siamo contro l'utero in affitto e contro chi promuove la maternità surrogata, soprattutto perché queste realtà calpestano i diritti delle donne. Per noi al primo posto c'è la tutela dei bambini: su questo punto, nel rispetto delle differenze, rivendichiamo con forza la nostra identità.

la bifobia è l'occasione per ribadire il nostro rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e dunque per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. non può che essere l'occasione per affermare il nostro doveroso e comune impegno a rispettare, proteggere e realizzare il pieno ed equo esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di lesbiche, *gay*, bisessuali, *transgender* e intersessuali. Colleghe e colleghi, questa più di altre è una ricorrenza che ha senso riempire di contenuto. È infatti innegabile che a diciotto anni dall'istituzione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, bifobia e la transfobia e a trentatré anni dalla storia data del 17 maggio 1990, quando l'omosessualità venne rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall'Organizzazione mondiale della sanità, c'è ancora tantissimo da fare. Orientamento di genere e identità sessuale sono ancora ai primi posti tra le cause di discriminazione negli spazi pubblici, sul luogo di lavoro e persino in famiglia. I discorsi d'odio sono un fenomeno endemico nel nostro Paese e non ci è concesso di abbassare la guardia. Si contano più di 2 miliardi di persone che vivono in Paesi in cui l'omosessualità è illegale. Per le giurisdizioni di 11 Paesi le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso sono ancora passibili di pena capitale. Se è innegabile che negli ultimi decenni si siano riscontrati segni di progresso a livello globale e siano stati fatti passi avanti anche nel nostro Paese - penso alle unioni civili, ad esempio è intollerabile che continuino ad essere consentite, talvolta legittimate discriminazioni ed esclusioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Abbiamo sottoscritto la mozione in discussione oggi perché riteniamo un fatto importante che unitamente il Senato prenda posizione contro discriminazioni che riteniamo del tutto intollerabili. Eppure - diciamolo chiaramente - questo testo prevede davvero il minimo sindacale e dispiace moltissimo constatare che il Parlamento, ancora una volta, dimostri di essere drammaticamente indietro rispetto al Paese. Non è forse ora di approvare finalmente una legge contro i crimini d'odio fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità? Non è forse pronto il nostro Paese per il matrimonio egualitario? Non è forse ora di riconoscere a singoli e coppie non etero il diritto di adottare? Non è forse ora di rivedere tutta la materia della fecondazione assistita e della gestazione per altri? Noi pensiamo di sì. Pensiamo che l'altro da noi, la diversità, costituisca sempre un arricchimento. Odio, disprezzo, discriminazioni, esclusione nei confronti di ciò che si ritiene diverso da sé altro non sono se non una forma di violenza che genera regressione e spinge verso fanatismi inaccettabili. Le discriminazioni e le parole d'odio pesano nella vita di tante, troppe persone, sono catene che le tengono legate senza dar loro la possibilità di esprimersi, di essere sé stesse, di contribuire alla vita sociale, culturale ed economica della nostra società. Non si può far finta di niente, colleghi. Non possiamo sminuire. Ricordiamo che le parole umiliano, legittimano la violenza e talvolta uccidono. E certi discorsi fatti di recente anche da autorevoli esponenti della maggioranza contribuiscono a creare il terreno, l'*humus* dentro il quale attecchiscono discriminazione e violenza. La ferita alla libertà della singola persona offende la libertà di tutti e purtroppo non sono pochi gli episodi di violenza morale e fisica che ogni giorno nel nostro Paese colpiscono la vittima, ma colpiscono anche tutte e tutti noi. Crediamo, invece, che sia indispensabile educare a una cultura della non discriminazione, perché il riconoscimento di ogni individualità è la base sulla quale si costruisce il nostro civile vivere collettivo. - badate bene - il rispetto dei diritti di ogni persona, l'uguaglianza tra tutti i cittadini sancita dalla nostra Costituzione e condivisa dagli ordinamenti internazionali che abbiamo fatto nostri non sono derogabili in nessun modo. A ribadirlo l'anno scorso per l'ennesima volta, di fronte ai numeri ancora terribili dei reati d'odio - accertati addirittura 1.445 - il presidente Mattarella. Questo Parlamento non può, non deve restare indietro: deve combattere la discriminazione e la violenza, i discorsi di odio basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Quanto a noi, continueremo a impegnarci per promuovere misure legali, politiche e finanziarie di lotta contro la discriminazione in cooperazione con la società civile. L'uguaglianza, il rispetto della dignità e il rispetto della diversità sono valori centrali, imprescindibili. Ciascuno dovrebbe liberamente poter essere sé stesso e amare chi ha scelto senza paura. Le attitudini personali e l'orientamento sessuale non possono costituire motivo per aggredire, schernire, negare il rispetto dovuto alla dignità umana, perché laddove ciò accade vengono minacciati i valori morali su cui si fonda la stessa convivenza democratica. È con l'auspicio che alle parole che sentiremo oggi possano seguire finalmente fatti concreti e provvedimenti giusti che noi di Alleanza Verdi e Sinistra voteremo a favore della mozione. signora Ministra, è molto positivo che tutti i Gruppi assieme sottoscrivano una mozione per impegnare il Governo a promuovere la depenalizzazione universale delle condotte relative ai rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso. Come spiegato bene nella mozione, ancora 71 Paesi, soprattutto arabi e africani, prevedono leggi punitive contro l'omosessualità. L'ultimo rapporto di Amnesty individua nelle violenze contro le persone LGBT una delle principali forme di violazione dei diritti umani, sia essa legata al piano giuridico, sia essa una forma di discriminazione culturalmente radicata e rafforzata da una politica di estrema destra. Non dobbiamo neppure uscire dai confini dell'Europa per osservare discriminazioni deliberate dall'alto: lo scorso anno, solo grazie alle grandi mobilitazioni internazionali e dell'opinione pubblica, in Ungheria non è passato il *referendum* sulla legge del Governo Orban che equiparava l'omosessualità alla pedofilia. In Polonia ancora oggi ben 79 unità amministrative si dichiarano zone libere dalle persone LGBT. Molte altre sono state costrette a ritirare la risoluzione solo dopo le pressioni della Commissione europea. Purtroppo, si tratta proprio dei Paesi di Visegrad, grandi amici del Governo italiano. Purtroppo anche questo Governo non è senza peccato. Discrimina le famiglie omogenitoriali, impedendo ai Comuni di iscrivere il genitore non biologico nel registro di stato civile. Una famiglia è composta da un padre e una madre, si continua a ripetere e l'abbiamo sentito oggi anche in quest'Aula, ma cos'è questa frase se non una discriminazione per le migliaia di coppie omosessuali con figli che vivono in Italia? *(Applausi)*. Soprattutto, è una discriminazione dei loro figli da parte di un Governo i cui esponenti sottolineano la loro straordinaria sensibilità ai temi dell'infanzia. Una discriminazione che la Corte costituzionale, già con sentenza n. 32 del 2021, aveva chiesto di l'Italia non ha ancora una legge che punisce l'istigazione all'odio contro gli omosessuali, una legge che è stata introdotta nella maggior parte dei Paesi europei europei e che è essenziale per offrire uno strumento di difesa nell'epoca in cui sui *social* *media* si animano vere e proprie campagne di istigazione all'odio e alla violenza contro le minoranze sessuali e le donne. Insomma, anche da noi ci sarebbe molto da fare. Oltre a chiedere in maniera unanime che l'omosessualità venga depenalizzata in tutto il mondo, una cosa che trovo assolutamente positiva, facciamo dei passi in avanti anche in Italia, dove tutto dipende da noi. Riprendiamo il disegno di legge contro l'omotransfobia facciamo finalmente un provvedimento che garantisca gli stessi diritti ai figli delle famiglie omogenitoriali.

per essere riusciti a mettere insieme una mozione unitaria e poter oggi, nella Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, prendere una posizione in cui il Parlamento chiede solennemente al Governo di fare una cosa importante, cioè di mettersi alla testa di quei Paesi che sono contro la criminalizzazione dell'omosessualità, della bisessualità e della transessualità in tutto il mondo e chiederne la depenalizzazione. Penso che sia un impegno importante che il Governo si assume assume e noi come Parlamento dovremmo pungolare il Governo in questa direzione e verificare che l'azione sia coerente con questo impegno. giustamente, la mozione che abbiamo sottoposto e che voteremo quest'oggi si dilunga moltissimo sulla situazione in Paesi come quelli dell'Africa o del Medio Oriente, dove le violazioni dei diritti umani si concentrano anche nei confronti delle persone omosessuali, con pene ovviamente contrarie all'umanità; sono pene degradanti, che che ripugnano a un Paese giuridicamente civile come il nostro. Tuttavia, non c'è soltanto un'omofobia di Stato nei Paesi africani come l'Uganda - abbiamo parlato della legge recentissima, del marzo 2023, quindi la situazione va anche peggiorando - o nel Medio Oriente. Esiste un'omofobia di Stato anche in Europa. Sappiamo bene, per esempio, che in Russia ci sono leggi molto pesanti e molto gravi che condannano quella che viene chiamata propaganda dell'omosessualità. Sappiamo che nell'Unione europea esistono Paesi, come l'Ungheria o come la Polonia,

costituirsi insieme ad altri Paesi davanti alla Corte di giustizia che aveva aperto una procedura di infrazione contro l'Ungheria. L'Italia, purtroppo, non si è unita ai Paesi che hanno sostenuto l'azione della Commissione europea. Penso che dopo la mozione di oggi questo chiaramente non accadrà più, Ministra. Tornando alla Russia, in quel Paese c'è addirittura chi, come il patriarca Kirill, dà la colpa della guerra e dell'invasione dell'Ucraina al fatto che nei Paesi occidentali - grazie al cielo e grazie alla democrazia e allo Stato di diritto - le persone omosessuali hanno diritto di vivere vivere libere, come lei ha detto, signora Ministra. Oggi è la giornata contro l'omofobia e noi dobbiamo, anche giustamente, in questa alta sede istituzionale, fare un po' i conti con la situazione del nostro Paese, dove quella libertà di cui lei ha parlato, signora Ministra, non è ancora conquistata pienamente. Abbiamo fatto un grande passo in avanti sulle unioni civili, che nel 2016, proprio in questi giorni di maggio fu approvata, e che è servita molto più di tante leggi penali per far passare l'idea nella società che una coppia di uomini o di donne che si amano vada celebrata nella nostra comunità come qualsiasi famiglia che nasce. Purtroppo, però, non abbiamo ancora completato quel tassello che ci manca e che ancora oggi ci fa stare in questo libro, nel rapporto di Amnesty International. Mi riferisco a una legge che condanni l'odio, la discriminazione e la violenza nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e trans. Glielo dice, signora Ministra, un parlamentare che non è un particolare particolare tifoso delle norme penali per risolvere le questioni; non penso sia quello lo strumento. Eppure, noi abbiamo nel nostro ordinamento l'articolo 604 del codice penale, che condanna la discriminazione, l'odio e la violenza per motivi etnici, religiosi, nazionali, razziali; quindi, il nostro ordinamento conosce le norme antidiscriminatorie, e non si capisce perché un pezzo del mondo, che pure soffre di discriminazioni storiche, non venga coperto esattamente dalla medesima legge e dal medesimo articolo 604 del codice penale. *(Applausi)*. Abbiamo perso una grande occasione nella scorsa legislatura per la sciagurata scelta di venire a contarci in quest'Aula quando sapevamo benissimo che non avevamo i numeri, perché non eravamo andati sotto di un voto a scrutinio palese nel mese di luglio e andare a ottobre a uno scrutinio segreto era un suicidio, forse voluto. Però, signora Ministra, mi aspetto di vedere quelle aperture

che è anche sicurezza, signora Ministra. Essere liberi per le persone LGBT significa anche vivere sicuri, e questa sicurezza ancora non l'abbiamo. Mi lasci dire un'altra cosa, e mi avvio alla conclusione. La libertà, quel concetto che ella, signora Ministra, ha evocato e che è caro al nostro cuore, non può esistere senza l'uguaglianza: si è liberi e uguali; non si può essere liberi e basta. Quindi l'omofobia va combattuta non soltanto quando è un cazzotto in un occhio mentre cammini per strada mano nella mano con il tuo compagno; l'omofobia non è soltanto la discriminazione sul lavoro o essere apostrofati per strada con parole volgari. Uguaglianza è anche sconfiggere per sempre l'idea, più diffusa di quanto non pensiamo, che le persone omosessuali sono meno delle persone eterosessuali, che sono per loro natura meno capaci e meno degne di accedere a certi istituti giuridici. Le faccio Le faccio un esempio: come è possibile che in tutta Europa e nei Paesi confinanti con l'Italia (la Slovenia, la Svizzera, la Francia) due persone omosessuali possono sposarsi e in Italia no? Qual è il concetto o l'idea per i quali noi scriviamo nella legge una discriminazione di diritto positivo, dicendo che certe persone non possono accedere a un istituto giuridico che è accessibile per loro in tutta l'Europa occidentale, nel Nord America, in molti Paesi del Sud America, ma in Italia no? Qual è la ragione e per quale motivo non siamo in strada a pretendere l'uguaglianza? Si dice: ma avete le unioni civili, di cosa vi lamentate?

nel mio sedile, non nel sedile di dietro. Quindi vanno bene le unioni civili, sono un bell'autobus; ma in quell'autobus noi stiamo seduti dietro. E questa cosa non può più durare, perché non esiste in Slovenia, non esiste in Francia, non esiste in Spagna, in Svezia, in Danimarca, in Islanda, in Gran Bretagna, in Germania (e smetto per carità di patria). *(Applausi)*. Ci aggiungo l'Argentina, per motivi che potranno ritornare utili. Questa dignità, questa capacità di accedere agli istituti giuridici vale anche per la filiazione: dire che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma è normalmente vero, ma non è vero se si dice che può vivere solo cresciuto da un papà e da una mamma, perché perché non esiste nessuno studio scientifico che lo confermi. La scienza non lo dice; questo è un luogo comune, non dissimile dal luogo comune che diceva che una persona bianca e una di colore non potevano sposarsi. Quel luogo comune faceva pensare che quella fosse la verità, cinquanta, negli Stati Uniti era impossibile. Oggi ripugna alla nostra coscienza, ma all'epoca sembrava normale. Le posso dire, signora Ministra, che forse tra vent'anni ci ripugnerà pensare che un tempo dicevamo che due omosessuali non potevano sposarsi o non potevano crescere sani dei figli, perché è contrario a quello che dice la scienza. È molto semplice. Allora, se vogliamo rimuovere l'omofobia di Stato, quella che uccide con la pena di morte, e se vogliamo rimuovere l'insicurezza di vivere in un Paese che ti tutela se sei ebreo, però se sei ebreo e *gay* ti tutela soltanto a metà, soltanto per la parte ebraica o soltanto per la parte di colore, soltanto per la parte della nazionalità, mentre per il resto puoi essere maltrattato, discriminato, picchiato e magari ucciso, quella parte lì va fissata. Ma ancor prima va stabilito un concetto preciso: uguali, signora Ministra, e dobbiamo tutti poter accedere a tutti gli istituti giuridici, senza nessuna eccezione, perché quella eccezione è il piccolo seme che fa nascere la grande omofobia.

Signora Presidente, oggi è uno di quei momenti in cui quest'Aula si presenta unita. Unita nel dire "no" in modo chiaro e netto all'omofobia e alle persecuzioni contro gli omosessuali attuate in alcuni Paesi africani, asiatici e mediorientali. Non possiamo che essere molto soddisfatti di essere riusciti ad esprimere una posizione unitaria di tutte le forze politiche, proprio nella Giornata internazionale contro l'omofobia. Con questa mozione dimostriamo che è possibile trovare un punto di incontro anche tra sensibilità e culture politiche diverse sui cosiddetti diritti civili; diamo al Paese il segnale che partiti lontani anni luce l'uno dall'altro sono in grado di avvicinarsi e camminare nella stessa direzione quando in ballo ci sono i diritti umani e la lotta a ogni genere di discriminazione. Le battaglie più importanti si vincono solo quando non ci sono divisioni, liti e scontri, perché questi danno un segnale di grande debolezza e finiscono per compromettere nobili cause che si vogliono sostenere. La mozione impegna, infatti, il Governo a partecipare alla costruzione di una coalizione dei Paesi che si impegna ad esercitare dovute pressioni nei confronti di quegli Stati che ancora considerano l'omosessualità un crimine o addirittura una malattia. Un impegno che noi di Forza Italia sentiamo profondamente in linea con i nostri valori, perché ha come suo presupposto uno dei principi cardine della concezione del mondo e della vita cristiana ed occidentale: il rispetto della persona umana, della sua dignità e della sua libertà individuale. Proprio oggi che si celebra la Giornata mondiale contro l'omofobia, è fondamentale ribadire, senza se e senza ma, che nessuno può essere discriminato o peggio perseguitato per le sue preferenze sessuali, per il suo modo di vivere l'affettività e la sessualità. La difesa del valore della persona, delle sue prerogative irrinunciabili e dei suoi diritti individuali universali e inalienabili si fonda sull'assunto, profondamente cristiano, che ognuno di noi, nella sua identità, è unico e irripetibile e che proprio per questo concorre ad arricchire, con le sue peculiarità, la grande famiglia umana. Difesa della persona, quindi, e dei diritti universali di ogni essere umano; promozione della libertà nello Stato di diritto e del buon senso. La nostra condanna all'omofobia, la nostra richiesta al Governo di contrastare i sistemi giuridici di quei Paesi che considerano l'omosessualità un crimine o una malattia si fonda sulla convinzione che in quegli Stati domina un'ideologia intollerabile, che vorrebbe eliminare un pezzo di realtà, negandola, perché non piace a chi comanda. Il fatto che la quasi totalità dei Paesi dove l'omosessualità viene perseguita si trovi al di fuori del Continente europeo non ci esime dal ricordare che, proprio noi europei, sappiamo bene cosa significa discriminare un pezzo di umanità in nome di una presunta società migliore. Il totalitarismo novecentesco nasce da questo tipo di assunto, dalla pretesa di sradicare il male, la malattia, vera o presunta, di sanare la società. La stessa repulsione per questo tipo di assunto ci spinge a difendere la famiglia naturale e ad opporci con tutte le nostre forze a nuove e pericolose ideologie totalitarie. Continueremo ad opporci a pratiche come l'utero in affitto, una pratica che umilia le donne, mercificando il loro corpo, così come riduce il bambino stesso ad oggetto di compravendita, aumentando un *business* umano che nulla ha a che fare con il progresso. Allo stesso modo ci opporremo all'introduzione, più o meno esplicita, dell'ideologia *gender* nelle scuole, perché la libertà educativa della famiglia rimane per noi al centro del rapporto tra i più piccoli e la sfera affettiva e sessuale. Impediremo degenerazioni come quella cui stiamo assistendo nel mondo anglosassone, che portano spesso operatori socio scolastici ad indurre negli adolescenti la prospettiva della transizione di genere, in alcuni Paesi addirittura senza il consenso genitoriale. Continueremo a sostenere, culturalmente, politicamente ed economicamente la famiglia naturale, cellula fondamentale della nostra società, così come riconosciuto dalla nostra Costituzione: non per limitare libertà e diritti di qualcuno, perché da liberali è una prospettiva che ci inorridisce, ma per garantire, attraverso di essa, la continuità della nostra società e la sostenibilità economica del nostro Paese e del nostro bilancio pubblico. La lotta all'omofobia è e deve essere sacrosanta. Noi di Forza Italia abbiamo sempre difeso la libertà di ciascuno. Attenzione, però, ad utilizzare l'omofobia come arma ideologica, dando dell'omofobo a chiunque voglia difendere, proteggere e tutelare la famiglia, il corpo della donna e i bambini. Il rischio è la banalizzazione e, quando si banalizza, si rischia di fare un regalo ai veri omofobi, che invece vanno puniti. di tale lotta il faro del dibattito politico, oggi ed ogni volta che discutiamo di diritti civili, evitando approcci di tipo ideologico, sono certa che eviteremo di spaccare la politica, la società italiana ed il Paese in fazioni contrapposte, così come avvenuto, purtroppo, con provvedimenti quali il disegno di legge Zan. Per tutte queste ragioni, il Gruppo Forza Italia al Senato voterà convintamente a favore di questa mozione.

sono sempre più drammatiche: è di poco fa, infatti, la nota stampa secondo cui ci sono 21 fiumi esondati in più punti, 22 corsi d'acqua che hanno superato il livello di guardia tre, che è il massimo allarme, sono aumentati a 35 i Comuni con allagamenti tra la Romagna e il bolognese. Purtroppo si contano in questo momento addirittura morti, sette in provincia di Forlì-Cesena e un uomo nel ravennate. Sembra davvero di trovarsi in un film apocalittico, distopico,

Però, colleghe e colleghi, non parliamo di vittime dell'alluvione, come pure ho sentito dire nel corso di questa giornata in quest'Aula, perché sono vittime della crisi climatica e, finché non ci uniremo tutti, magari come stiamo facendo per la mozione in discussione, per mettere in campo davvero ogni azione possibile, magari anche quelle che adesso sembrano impossibili, per riportare indietro le lancette di questa crisi, nessuno di noi potrà dirsi esente da responsabilità. *(Applausi)*. Le parole di cordoglio e di vicinanza sono naturalmente doverose, ma agire sul serio, con coraggio e con serenità non è più rinviabile. I nostri giovani ci implorano.

dei disturbi mentali, chiarendo così una volta per tutte che non si tratta di nessuna devianza e tantomeno di nessuna patologia e che l'orientamento sessuale fa semplicemente parte dell'identità di ciascuno di noi, di ciascun essere umano. C'è tuttavia un altro anniversario che ricorre quest'anno, meno noto, ma forse addirittura più importante. Oggi sono infatti cinquant'anni da quando nel 1973 l'Associazione americana degli psichiatri rimosse l'omosessualità dal DSM, il manuale diagnostico e statistico allora più autorevole del mondo. Fino a quel momento l'omosessualità era considerata un disturbo sociopatico della personalità e veniva curato di conseguenza: succedeva nel cuore dell'Occidente, sia in Europa che negli Stati Uniti. Le persone LGBT non solo erano legalmente perseguitate, ma venivano sottoposte ad ogni specie di vera e propria tortura: castrazioni, lobotomie e sedute psicanalitiche di conversione dell'orientamento sessuale sono state effettuate su migliaia e migliaia di uomini e donne in Europa e negli Stati Uniti, ancora fino agli anni Settanta dello scorso secolo.

convertire l'omosessualità, che l'omosessualità si cambia, si cura: si tratta delle cosiddette teorie riparative, una recrudescenza di barbarie antiscientifica, che va respinta con forza e decisione e che infatti in alcuni Paesi è esplicitamente fuori legge e speriamo che possa essere messa fuori legge presto anche in Italia. Appare inoltre certamente superfluo ricordare in quest'Aula come *gay*, lesbiche e in generale le persone non conformi furono tra le vittime obiettivo della follia nazifascista, che le ha perseguitate e rinchiuse nei *lager* e spedite al confino per via del loro modo di essere. È quindi da quel 1973 che per la prima volta si aprì una vera crepa in questa visione assurda e l'omosessualità smise di essere considerata una patologia. Tutto iniziò da lì. È infatti a partire dagli anni Settanta che i movimenti LGBT hanno intrapreso una marcia per affermare i propri diritti, innanzitutto il diritto alla libertà di essere se stessi. Questa marcia ha visto naturalmente alterne fortune. Così, mentre i diritti come l'accesso al matrimonio, la filiazione, il riconoscimento dei figli, leggi specifiche a tutela contro l'odio e la discriminazione transfobiche sono realtà in molti Paesi del mondo, in ben 71 Paesi invece - e sottolineo che sono aumentati di recente, quindi c'è una recrudescenza dell'odio verso le persone LGBT - l'omosessualità è punita finanche con la pena di morte, la flagellazione, la lapidazione l'impiccagione, come abbiamo più volte ricordato in quest'Aula. Ecco perché è importante questo voto di oggi ed ecco perché è così importante che sia unitario. È vero, possiamo pensarla in maniera diversa su tante cose, addirittura su tutto, ma tutti noi non possiamo che essere d'accordo e riconoscere che il diritto alla vita, all'integrità fisica e psicologica, la libertà e la dignità della persona umana sono valori supremi e inviolabili *(Applausi)*, che non possono non possono soggiacere a nessun altro tipo di considerazione. Certamente non possono soggiacere ad eventuali valutazioni di consenso politico. Tengo a ricordare oggi anche un'altra cosa in quest'Aula che sta per votare un impegno così importante a questo Governo; una legge che in pochi ricordano, ma che è stata fondamentale. Si tratta della legge n. 13 del 2007 che, all'articolo 12, reca una norma meglio nota come norma Grillini-Silvestri, dal nome dei proponenti. Dalla sua entrata in vigore nel 2007 tale norma ha contribuito a salvare ben 15.000 persone. Persone che probabilmente avrebbero trovato la morte o il carcere nei loro Paesi di origine a causa del loro orientamento sessuale. Come italiane e italiani dobbiamo essere orgogliosi di questa legge e sarebbe una follia metterla in discussione, tanto più oggi. oggi. La persecuzione nel mondo delle persone LGBT non si è infatti affatto fermata come abbiamo sentito, anzi. L'International gay and lesbian association (ILGA), un'associazione "ombrello" che riunisce oltre 400 associazioni mondiali e che è membro osservatore presso le Nazioni Unite, nel recente rapporto annuale denuncia proprio la recrudescenza dei fenomeni di odio verso le persone LGBT: ci ricorda come la stessa Europa non ne sia purtroppo esente, citando in particolare i due attacchi terroristici avvenuti nel 2022 fuori dai locali frequentati dalla comunità LGBT, in Norvegia e in Slovacchia, dove sono rimaste ferite 22 persone e uccise 4 persone. Diciamo da anni che l'incitamento all'odio in tutte le sue forme si traduce in violenza fisica reale, ha commentato la direttrice esecutiva di ILGA Europe Evelyne Paradis, alla pubblicazione dell'indagine annuale. Anche il nostro capo dello Stato Mattarella oggi ha voluto far sentire la sua voce. «Omofobia, bifobia e transfobia costituiscono un'insopportabile piaga sociale ancora presente e e causa di inaccettabili discriminazioni e violenze, in alcune aree del mondo persino legittimate da norme che calpestano i diritti della persona», ha affermato il presidente Mattarella. Dal 2007 quando venne istituita dal Parlamento europeo la Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, la sensibilità della coscienza collettiva verso questi temi si è accentuata. L'azione di contrasto di numerosi episodi di violenza che la cronaca continua a registrare non può cessare. Contro le manifestazioni di intolleranza dettate dal misconoscimento del valore di ogni persona deve venire una risposta di condanna unanime. È compito delle istituzioni elaborare efficaci strategie di prevenzione che educhino al rispetto della diversità dell'altro e all'inclusione. Quindi oggi noi

anche l'auspicio delle associazioni LGBT, che da sempre chiedono impegni concreti nel contrastare odio e discriminazione e hanno seguito la nascita e l'evoluzione di questa mozione fin dall'inizio. A tutte e tutti loro, da sempre impegnati per rendere il nostro Paese più accogliente e giusto, va il mio ringraziamento per il lavoro instancabile e per il loro sostegno. Sto per terminare, signor Presidente. In conclusione, ci tengo a ringraziare una persona speciale, Franco Grillini *(Applausi)*, che è un monumento vivente della lotta per i diritti e la libertà nel nostro Paese, per aver sostenuto fin dal primo momento l'idea che questa mozione dovesse essere unitaria. Nel corso delle conversazioni in cui ne abbiamo parlato mi ha detto: ma guarda che quelli là li ammazzano veramente, mica per scherzo; noi dobbiamo fare qualcosa di concreto, basta belle parole. Questo lo ha detto non con questo accento, ma con il suo bell'accento bolognese, verace ed elegante al tempo stesso. Con Con questo voto consegniamo in maniera unitaria nelle mani del Governo un impegno concreto, affinché l'Italia si faccia promotrice in tutte le sedi istituzionali europee ed internazionali della cessazione della criminalizzazione delle persone LGBT nel mondo, che vengono perseguitate per la sola legittima aspirazione di essere se stesse e di essere libere di amare chi sentono di amare. Confidiamo che il Governo prenda questo impegno seriamente, come merita, e faccia dell'Italia il Paese capofila per la decriminalizzazione dell'omosessualità nel mondo.

Signor Presidente, come Gruppo Lega noi abbiamo aderito e firmato questa mozione per due ragioni. Innanzitutto, perché mettere mettere in evidenza che non esistono nessuna devianza e nessuna patologia, ma che l'orientamento sessuale fa semplicemente parte dell'identità di ogni essere umano penso che ormai sia una questione che hanno capito e sanno tutti, ed è sicuramente un segnale di progresso e di civiltà. modo, sappiamo che, essendoci 71 Paesi al mondo che hanno leggi punitive contro l'omosessualità e gli orientamenti sessuali, è giusto mobilitare a livello internazionale tutti gli Stati per fare in modo che si promuova una vera e propria depenalizzazione, laddove effettivamente ancora ci sono norme che non tengono conto dei diritti umani universali delle persone. Abbiamo sottoscritto e portato avanti questa mozione anche perché abbiamo lasciato fuori l'ideologia; abbiamo lasciato fuori alcune ideologie che sono portate avanti anche da alcuni movimenti, come quello LGBTQI. È vero che ci sono alcune questioni che vengono portate avanti e su cui noi non siamo assolutamente d'accordo. d'accordo. Abbiamo tenuto fuori le ideologie: giusto e corretto, perché solo così ci può essere un atteggiamento costruttivo tra maggioranza e opposizione su questi temi. Ci sono uomini che amano altri uomini o donne che amano altre donne?

che a mio figlio venga insegnato il rispetto per le persone, non solo per l'orientamento sessuale che hanno, ma anche per il sesso, per la religione, per l'etnia, per le convinzioni politiche e per la libertà di espressione, che spesso e volentieri purtroppo non viene garantita. Rispetto per la persona significa anche rispetto per le differenze. Purtroppo oggi si è un po' allergici al discorso della differenza, in tanti casi perché si pensa che significhi esclusione. differenze per noi sono considerate una ricchezza e vanno assolutamente valorizzate: questo è l'insegnamento che dobbiamo portare nelle scuole. cosa ci ha spinto a dire che questa è la strada giusta purché si lascino fuori le ideologie? A quali ideologie facciamo riferimento? A quelle che invece vogliono imporre una sorta di modello nella nostra società; quelle che vogliono indottrinare i nostri figli *(Applausi)*; quelle che impongono sostanzialmente una propaganda, una manipolazione. Con tutto il rispetto, dobbiamo lasciare ai nostri figli il tempo di maturare consapevolmente le loro scelte; invece purtroppo ci sono alcune ideologie, anche nell'Unione europea, che pretendono che i minori vengano trattati come adulti, specialmente nella sfera sessuale, e noi su questo non siamo d'accordo. Proprio per questo riconosciamo e assolutamente condividiamo il fatto che il Governo non abbia aderito a quell'iniziativa che alcuni Paesi europei hanno preso nei confronti dell'Ungheria e della Polonia. Si possono tutelare benissimo i diritti individuali.

Tener fuori le ideologie significa che si possono benissimo tutelare i diritti individuali senza per questo distruggere la famiglia. *(Applausi)*. In alcuni casi che la famiglia naturale non esiste, che è una pura invenzione nostra. Peccato che l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani recita, al comma 2, che la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Tenere fuori le ideologie significa non riconoscere la teoria *gender.* Ci sono casi di disforia di genere? Sì, giustamente

di perdere l'identità, cosa che potrebbe essere devastante, perché anziché vivere ogni giorno chi si vuole essere, noi diciamo che bisogna vivere ogni giorno chi davvero si è. Questo vuol dire rafforzare l'identità

diventare diritti, come per esempio la pratica della maternità surrogata o l'utero in affitto. Insomma, alla fine selezionare ovociti sui cataloghi mi ricorda una pratica un po' razzista*,* mentre giustamente dobbiamo sempre combattere il razzismo. modo, va affermato il diritto delle donne a non essere sfruttate come strumenti di procreazione: anche questo è un altro diritto che va affermato. *(Applausi).* Se teniamo fuori

Lasciando perdere le ideologie, possiamo assolutamente aumentare le pene nei confronti di chi discrimina, non solo per etnia, sesso o religione, ma inserendo anche l'orientamento sessuale, però lasciando fuori le ideologie. Signor Presidente, colleghe e colleghi, Ministra, poco più di trent'anni ci separano dal giorno in cui l'Organizzazione mondiale della sanità rimosse l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Il 17 maggio è una giornata storica e non potevamo permettere che passasse nel silenzio delle Aule parlamentari, né che anche da questi luoghi non si alzasse una voce contro ogni forma di violenza legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Sarebbe stata un'afasia insostenibile di fronte a quanto c'è ancora da fare contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Nel mondo - è vero - li uccidono veramente, ma anche da noi. Oggi il Presidente della Repubblica ci ha richiamati a una risposta unanime. Solo ieri ci aveva preoccupati il ritardo per cui il ministro Valditara Valditara non aveva ancora emanato la consueta circolare che richiama l'importanza di celebrare, e dare risalto, alla Giornata internazionale contro l'omotransfobia come mezzo per diffondere nelle generazioni più giovani una cultura dell'uguaglianza e del rispetto delle differenze e dell'inclusione. Sempre il presidente Mattarella ha richiamato efficaci strategie di prevenzione che educhino al rispetto della diversità dell'altro e all'inclusione. Sono questi i progetti contro gli stereotipi di genere che si fanno nelle scuole di ogni ordine e grado, nulla a che vedere con fantomatiche ideologie *gender* e con l'indottrinamento di bambine e bambini. Sono questi i progetti che tanto vi spaventano. Non abbiamo inteso comunque, per la gravità della battaglia che dobbiamo fare, pregiudicare un percorso unitario, che vede oggi il Senato approvare all'unanimità la mozione presentata dalla collega Maiorino, una cornice condivisa, come dovrebbero essere le battaglie su questi temi e sui diritti universali. però, è scivolata al trentaquattresimo posto nella lista dei Paesi europei per la tutela dei diritti delle persone LGBTQI+. questo dibattito avviene in un momento caratterizzato da un attacco senza precedenti alla cittadinanza di queste persone, un attacco culturale e politico, già fortemente stigmatizzato in sede europea da ben due risoluzioni del Parlamento di Strasburgo nelle ultime settimane: condanna di diffusione di retorica anti-diritti, anti-*gender* e anti-LGBT, condanna che ci accomuna a Paesi come l'Ungheria e la Polonia. *(Applausi)*. Io non voglio e sono preoccupata per il mio Paese, se viene accomunato su questi temi a Paesi come l'Ungheria e la Polonia. Oggi però può essere un giorno di riscatto per noi. Non possiamo non dire, perché lo votiamo, che anche in questo testo avremmo preferito leggere "identità di genere", perché c'è una specificità che riguarda la dignità delle persone *trans*, che nei Paesi che noi condanniamo con questa mozione sono quelle ancora più perseguitate, che ha diritto di essere riconosciuta, perché, come ci ha ricordato la Ministra, è nel corpo che la libertà si fa sostanza e quel corpo, quell'orientamento e quell'identità di genere che le persone vivono devono essere rispettati. Proprio in questi giorni è in libreria un testo che si intitola «Indietro non si torna»: è la storia di Monica Romano, consigliera comunale di Milano, una lettura che consiglio. Ebbene, Monica Romano, ripercorrendo la sua vicenda e la differenza tra le battaglie degli anni Novanta e oggi l'odio è strisciante, nascosto e difficilmente decifrabile; si annida tra le parole e i silenzi, celandosi dietro l'ombra di una spaventosa ipocrisia. Quanta ipocrisia su questi temi, colleghe e colleghi, dobbiamo combattere in questo Paese. *(Applausi)*. Oggi tutti insieme con questo testo condanniamo i Paesi che criminalizzano l'omosessualità in Africa e altrove. È una scelta importante, a cui dobbiamo far seguire conseguenze. Alcuni di questi Paesi - in particolare Nigeria, Gambia, Tunisia, Algeria, Marocco, Senegal e Ghana - sono attualmente ancora considerati di origine sicura ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, con la conseguenza che che la domanda può essere rigettata con procedura accelerata, se il richiedente non dimostra la sussistenza di gravi motivi per far ritenere superata la presunzione di sicurezza del Paese di origine. Insieme oggi decidiamo di far seguire a quest'approvazione un cambio di passo da parte del Governo sul riconoscimento di questi Paesi: non è a questo che serve una mozione siffatta? Del resto noi siamo un Paese dell'Unione europea, che si è dotata di un'importante strategia LGBT, sin dal 2019, dalla Commissione von der Leyen. Sulla dignità di queste persone e sul riconoscimento e sulla tutela dei loro diritti si gioca una parte importante della nostra partecipazione a testa alta al processo di integrazione europea, un'Europa inclusiva e della cittadinanza. Eppure, contro quell'Europa solo qualche settimana fa si è scelto qui di alzare un muro, dando un parere negativo al regolamento relativo al certificato europeo di filiazione. *(Applausi)*. Vedete, colleghi, non dovremmo dividerci su queste questioni, perché davvero non parliamo di ideologia, ma di persone, della loro dignità e della loro cittadinanza. La dignità delle persone, di tutte le persone, non può essere frammentata, accogliendone solo alcuni aspetti: la dignità o è intera o non c'è; o si riconosce la dignità di persone *(Applausi)*, di lavoratrici e lavoratori, di persone che hanno figli e fanno famiglia (perché esistono le famiglie, non i modelli astratti persone discriminate, oggetto di violenza, come le persone trans, e dei percorsi faticosissimi - altro che moda, altro che capricci! *(Applausi)* - che devono attraversare per affermare la loro identità ad esempio le studentesse e gli studenti che chiedono le carriere *alias*. O si riconosce la pari dignità di cittadine e cittadini o, molto semplicemente, si continua a discriminarli e renderli invisibili, privandoli di elementari diritti. trent'anni fa, nel 1993, questo Paese si dotò della legge Mancino, contro i discorsi d'odio e le discriminazioni per motivi razziali. Già allora, Franco Grillini, di cui tutti noi riconosciamo il protagonismo contro questi fenomeni, aveva proposto che quella legge si occupasse anche di omofobia, ma non si fece una scelta per farla approvare.

Vedete, colleghi, il Partito democratico voterà a favore di questa mozione per l'impegno a livello internazionale e perché speriamo che segni davvero un cambio di passo,

ritengo che sia di assoluta importanza una riflessione sul fatto che, da un lato, solamente dal 1990 ci si sia liberati da un concetto che sembra riportare agli oscuri pregiudizi medievali e, dall'altro, ci siano tante Nazioni che ancora oggi non solo non condividono quanto affermato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 1990, trentatré anni fa, ma anzi promulgano, emanano e soprattutto applicano leggi che hanno orientamento esattamente opposto. lungo infatti l'elenco di Paesi dove ancora esiste la punizione, anche estrema, per reati riconducibili all'orientamento sessuale. L'Occidente e i Paesi evoluti, economicamente molto evoluti e dominanti, devono altresì riflettere sul perché ancora oggi si possa osservare passivamente la triste evoluzione regressiva che permane in così tanti luoghi: senza che la comunità internazionale muova passi concreti, e non fittizi, verso investimenti che sostengano politiche ed iniziative di aiuto e cooperazione volte a emancipare socialmente, economicamente e culturalmente i popoli che ancora subiscono violenze fisiche e psicologiche. Ci si deve indignare di questo oggi, perché questo è il tema che stiamo veramente affrontando. Tuttavia, lo stesso va inquadrato in una più ampia visione di limitazioni o privazioni dei più elementari diritti di libertà, di azione e di pensiero, sia per quanto riguarda gli orientamenti sessuali sia per quello che concerne gli orientamenti religiosi, politici o sociali. Si consolida sempre più la spiacevole sensazione che convenga a qualcuno lasciare quei popoli nell'oppressione e nell'ignoranza, per poter gestire - con il tiranno di turno - le innumerevoli risorse naturali che albergano in quei luoghi o qualsiasi altro interesse superiore, che a tutto risponde tranne che al rispetto della dignità delle persone che vivono in quei Paesi, che sono vittime delle oppressioni. Il 17 maggio sia pertanto un giorno di denuncia per tutto ciò che sottende a questa innaturale privazione di libertà per quanto attiene agli orientamenti sessuali, ma lo sia anche e soprattutto per mantenere alta l'attenzione e rilanciare la denuncia del complessivo quadro di abusi e vessazioni che vengono commessi in troppe parti del mondo, nel silenzio degli organismi internazionali. Su tutto questo noi di Fratelli d'Italia non saremo mai silenti e saremo sempre dalla parte di tutti coloro che sono soggetti a discriminazioni, abusi, pregiudizi e violenza per le loro presunte diversità, senza preconcetti, senza un pensiero unico e lasciando da parte qualsiasi ideologia; senza demonizzare la famiglia tradizionale, come avete citato poco fa, a fronte proprio delle formazioni sociali di cui si parlava poc'anzi. *(Applausi)*. È per questo che siamo favorevoli alla mozione.

Ne ha facoltà. ALOISIO *(M5S)*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'autonomia differenziata è lo strumento inventato dalle Regioni più ricche per tentare di tenersi quasi interamente l'importo delle tasse che spettano allo Stato. Il provvedimento vide il proprio *incipit* nel 2001, quando, al termine dei lavori della bicamerale voluta da D'Alema e Berlusconi, si riformò il Titolo V della Costituzione. Successivamente, il 28 febbraio 2018, il Governo Gentiloni approvò tre accordi preliminari con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. C'è da chiedersi come mai, a soli quattro giorni dalle successive elezioni, un Governo che avrebbe dovuto occuparsi solo di ordinaria amministrazione abbia approvato accordi destinati a cambiare per sempre le sorti del Paese. Così arriviamo ai giorni nostri. Queste tre Regioni pretendono di gestire finanziamenti e competenze, circa duecento, secondo alcuni costituzionalisti, ma sono tre le materie più dedicate: sanità, scuola e infrastrutture e trasporti. Fortunatamente, a smontare le mire leghiste sul capitolo scuola è intervenuto proprio l'attuale Ministero dell'istruzione, secondo cui il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti è una prerogativa statale, che non può essere ceduta alle Regioni. Una posizione analoga sul capitolo sanità è poi arrivata dall'ordine dei medici, secondo cui l'autonomia aumenterà le diseguaglianze nella qualità delle prestazioni e negli accessi alle cure sanitarie. Infine, anche Confindustria ha preso una posizione netta contro questo provvedimento, che secondo il presidente dell'Unione industriali di Napoli, Jannotti Pecci, spaccherà in due il Paese, anche in considerazione della forte sperequazione infrastrutturale e dei trasporti. Onorevoli colleghi, cosa ancor più grave, si giustifica il trasferimento dei fondi facendo leva sul concetto di residuo fiscale, secondo cui la spesa per i servizi ai cittadini dovrebbe essere proporzionata alla capacità fiscale. Come dire che l'assistenza sanitaria e la scuola non devono essere le stesse per tutti, ma parametrate alla ricchezza del territorio. Si dice anche che questo provvedimento aiuterà il Sud, ma è quanto di più falso (questo lo dice soprattutto il ministro Calderoli). Secondo uno studio effettuato dal presidente della Svimez, Adriano Giannola, la Lombardia beneficerà di 106 miliardi in più, il Veneto di 41 e l'Emilia-Romagna di 43. Verranno penalizzate anche altre Regioni. Ricordo che sono ben quattro quelle settentrionali, che ricevono più di quanto danno e che sono tecnicamente assistite: Liguria,

la nostra Costituzione colloca in posizione di supremazia il diritto comunitario rispetto alla legislazione nazionale e proprio il Trattato della Unione europea reca l'obiettivo di rimuovere i divari territoriali tra gli Stati membri. non appena si profileranno condizioni di squilibrio territoriale, è lecito attendersi un pronto intervento della Corte costituzionale, che auspico possa fermare questa legge, destinata alla censura di incostituzionalità. Il MoVimento 5 Stelle dice no allo spezzatino dell'Italia. Do notizia all'Assemblea del fatto che la 7a Commissione permanente non ha ancora concluso l'esame del disegno di legge n. 551, recante «Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti».